La seduta è aperta *(ore 9,33).* Ricordo che nella seduta di ieri non si è proceduto all'approvazione del processo verbale della seduta del 7 dicembre. Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta di ieri,

Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta di ieri, occorre approvare il processo verbale della seduta del 7 dicembre.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca: «Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri». Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gentiloni Silveri, ha consegnato il testo delle dichiarazioni programmatiche rese alla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà. voglio dirlo subito: noi di Sinistra Italiana non daremo la fiducia a questo Governo; non la daremo perché

figuriamoci cosa stava succedendo nel Paese.

Chi non ha interesse ad ascoltare gli interventi in discussione generale è pregato di lasciare l'Aula; altrimenti vi invito a tenere un comportamento che consenta quanto meno di ascoltare

non ha nulla a che fare con il mondo reale, con quello che stava realmente accadendo nel mondo del lavoro. Più volte ho cercato, sia in Commissione lavoro che in quest'Assemblea, di evidenziare quello che stava realmente succedendo, ma questo Governo è stato assente. Ora, dopo questa bocciatura, voglio ricordare voglio ricordare che 20 milioni di italiani hanno detto no a questo Governo e allo scempio che si voleva fare della Carta costituzionale.

devastanti per la democrazia del nostro Paese e per il mondo del lavoro. Adesso chiedo a tutte le forze che hanno detto che volevano salvaguardare la democrazia di questo Paese

*(CoR)*. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, questa mattina ho letto un articolo di Staino sull'Unità dedicato alle prospettive del Governo e del partito. A un certo punto si cita un appuntamento programmatico in parte evocato anche nel dibattito di ieri (Taormina a maggio) e si dice che sia uno smacco per l'Italia che in quella occasione ci sia Gentiloni Silveri e non Renzi.

beffardo, velleitario e ricattatorio, quello che è avvenuto in Europa tra Ventotene (eravamo alla fine di agosto) e

aver confrontato le posizioni dell'Italia tra Ventotene e Bratislava - distanti non più di sei settimane e mezzo - francamente considero umilianti per un Paese fondatore dell'idea d'Europa assumere posizioni ricattatorie. Ecco perché il nostro Gruppo non ha particolarmente apprezzato - anche se comprende e li ritiene legittimi e comprensibili - i suoi richiami di ieri alla continuità con il precedente Esecutivo. Noi, però, in quest'Assemblea, per quanto concerne l'istituzione del Governo in Parlamento (perché ci sono un'istituzione «Governo» e un'istituzione «Parlamento» e, in democrazia, anche un'istituzione «Governo in Parlamento») ci aspettiamo dal suo Esecutivo un ripristino di lealtà e correttezza costituzionale, che sono cadute francamente in desuetudine rispetto all'abitudine ricorrente e sistematica al decreto-legge e al voto di fiducia, addirittura preventivo rispetto alla discussione generale. Ci aspettiamo, quindi, una forte discontinuità. Sotto questo profilo - mi consenta di dirglielo con tutta l'amabilità di cui la nostra tradizione politica è portatrice nelle sue dichiarazioni programmatiche lei ha fatto riferimenti solo indiretti alla consultazione referendaria di domenica 4 Sotto il profilo della correttezza istituzionale credo che questo sia un atto di disattenzione e in qualche modo di irresponsabilità. Non lo dico per far valere le ragioni, che hanno prevalso, del no rispetto al sì. Ma lei doveva perlomeno notare che in quell'occasione la partecipazione democratica, di cui parlava con tanta foga il collega che mi ha preceduto, è stata di un terzo maggiore rispetto a quella di tre mesi fa, nelle consultazioni amministrative per il tanto amato dagli italiani sindaco eletto. Questo deve essere un motivo di riflessione per tutti; lei non può eluderlo in nome di una continuità Io mi permetto di dirle che noi, piccolo Gruppo di opposizione (ma profondamente affezionato all'idea del costituzionalismo), riteniamo che quel 70 per cento M, Id, E-E, MPL)).* E in questo senso presenterò con molti colleghi del mio Gruppo (ovviamente aperta anche ad altri) l'immediata proposta di un'Assemblea costituente, un'Assemblea costituente nella quale, forti dell'esperienza che abbiamo vissuto qui in quest'Aula, il parere del Governo possa essere richiesto dall'Assemblea, ma non si possa fare una riforma costituzionale firmata e targata dall'Esecutivo. La Costituzione è un atto che vincola i cittadini, il Parlamento e il Governo. Non può votarsi una riforma costituzionale tutta quanta del Governo, addirittura nominando il testo del Governo come testo di riferimento Noi ci auguriamo, per quegli impegni che ci attendono su questa materia ai confini tra la politica e la politica costituzionale, di poter ragionare pacatamente e di poter fornire il nostro contributo, critico ma appassionato. A proposito di passione, mi consenta un'ultima considerazione: quando lei era Ministro degli affari esteri le capitò di essere schiaffeggiato (a mezzo stampa, non secondo il codice Gelli) dall'allora Presidente del Consiglio per le posizioni che la Farnesina aveva assunto in materia di rapporti con Israele. In seguito (mi pare che il presidente Renzi abbia parlato di pilota automatico) ci siamo trovati nell'UNESCO al fianco

Sono cose di cui abbiamo disgusto. Avrei avuto piacere che, sia al momento del passaggio delle consegne con il presidente Alfano sia due mesi fa, invece che a mezzo stampa e per intervista, lei fosse venuto

Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio, con la riforma costituzionale pasticciata, pessima e pericolosa imposta al Parlamento dalla coppia Renzi-Boschi, coppia ancora ben inchiodata sulla tolda di comando, si è tentato di perpetrare un imbroglio agli italiani, ben nascosto da un quesito ingannevole che sbandierava tagli di poltrone e risparmi inesistenti, ma 20 milioni di italiani, accorsi in massa alle urne, hanno sventato la trappola e vi hanno sonoramente bocciati. Bocciati perché volevate togliere il diritto di voto, con l'obiettivo di allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni. Bocciati perché volevate togliere competenze, poteri e risorse alle Regioni ordinarie e passarli all'inefficiente Stato centrale. Bocciati perché milioni di italiani non hanno voluto vendere la propria libertà per un *bonus* o per una manciata di euro promessi da Renzi, perché questi italiani hanno voluto continuare ad essere donne e uomini liberi e padroni del proprio futuro e hanno capito il rischio di cedere sovranità del Paese all'Europa, alle banche e alla grande finanza. Bocciati soprattutto perché hanno voluto liberarsi di Renzi e del renzismo, che hanno già fatto troppi danni, oltre alla spaccatura del Paese che ha creato la campagna referendaria. Il Governo Renzi e Renzi, nonostante ciò che lui dica nei vari saluti di arrivederci e non di addio (come aveva promesso), lascia in eredità risultati pessimi. Segnalo l'alta disoccupazione, soprattutto tra i giovani, nonostante i 20 miliardi spesi in incentivi per le assunzioni che hanno drogato il mercato del lavoro. Segnalo la fuga di italiani all'estero (107.000 nel 2005), tra cui e soprattutto molti giovani qualificati. Segnalo il *record* storico di italiani in povertà assoluta: 4,6 milioni è il dato degli ultimi giorni confortato e ulteriormente irrobustito dall'aggiornamento che il 30 per cento degli italiani sono sulla soglia della povertà e, in particolare, le famiglie numerose monoreddito, con tre o più figli, che stanno aspettando ancora gli 80 euro promessi da Renzi nel 2014. Segnalo le tasse che non sono assolutamente diminuite. Segnalo l'aumento del debito pubblico di 105 miliardi, in media 105 milioni al giorno, solo per la spesa corrente. infatti, fosse aumentato il debito pubblico per gli investimenti: no, sono diminuiti sensibilmente ed anche la nuova legge di bilancio, approvata in fretta e furia, segnala per il 2017 un'ulteriore diminuzione dell'8 Che dire poi delle varie riforme pessime e devastanti come il *jobs act*, la buona scuola, la cosiddetta legge Delrio e il salva banche? Le faccio alcune domande, primo ministro Gentiloni. Pensando a Trump, che negli ultimi giorni ha assunto decisioni importanti sugli F35 o sul nuovo Air Force One, ordinato da Obama, di cui pare voglia cancellare ovvero ridimensionare l'ordine, lei cosa intende fare dell'aereo blu, il giocattolino acquistato in *leasing* da Renzi

pagando elevati costi di affitto e con un impegno enorme del personale del 31° stormo. Cosa intende fare con le Province, che sono al collasso per la scelta scellerata della cosiddetta legge Delrio e che ora, per effetto della bocciatura della riforma, restano in vita senza soldi, con la competenza sulle strade e sulle scuole? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Cosa intende fare con le scelte irresponsabili fatte dal Governo e dal ministro Padoan con la delega fiscale che, contrariamente all'obiettivo della semplificazione, ha introdotto un eccesso di adempimenti e le comunicazioni trimestrali dell'IVA? Lei, come Monti, che ha istituito il Ministero per la coesione territoriale, intende proseguire come Renzi favorendo oppure contrastando il più becero clientelismo, come quello fatto nei giorni scorsi con le promesse al governatore D'Alfonso in Abruzzo o a De Luca in Campania, che si è visto regalare 600 milioni per sanare l'ennesimo buco di bilancio? E che dire dell'immigrazione scellerata? Oltre 175.000 sbarchi, il 6 per cento in più rispetto al 2014; nessun rimpatrio. *Premier* Gentiloni, non fate controlli alle frontiere; lo sa lei che dei quasi 13.000 pakistani che hanno richiesto asilo, solo il 20 per cento è entrato via mare e l'80 per cento è entrato via terra, dalla Slovenia e dall'Austria, senza controlli? È per questo motivo che il pessimo Alfano, sul fronte anche dell'accoglienza che sta esplodendo, ha voluto lasciare il Viminale. Altro che «il Paese è in condizioni di maggiore sicurezza!». Il ministro Alfano lo chieda agli italiani che vivono interamente

rivendicando la propria sovranità, come recita l'articolo 1 della Costituzione. La Lega Nord, *premier* Gentiloni Silveri, farà in Parlamento, da qui in avanti, un'opposizione durissima e senza sconti al suo Governo

le dimissioni di Matteo Renzi sono venute dalla consapevolezza che la maggioranza che ha sostenuto il suo Governo ha visto bocciare dai cittadini quella riforma costituzionale che era insieme ragione e obiettivo del Governo e della legislatura. Il *referendum* cancella una riforma che io continuo a pensare fosse necessaria per il Paese ma, al di là delle caricature di questi giorni e delle cose che ho sentito anche già stamattina, quel *referendum* non cancella le tante riforme e il lavoro fatto in questi mille giorni. Abbiamo fatto cose utili per il Paese e per tanti cittadini; ne parleremo e le racconteremo nei prossimi giorni, leggeremo i risultati quando ci sarà la serenità e la possibilità di farlo. Lei oggi, presidente Gentiloni Silveri, con il suo Governo e la sua maggioranza si assume con coraggio una responsabilità non semplice: portare il Paese alle elezioni affrontando questione urgenti per il Paese stesso, per l'Italia, come intervenire sul sistema bancario, consolidare il lavoro iniziato per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, affrontare impegni internazionali (compreso il tema del governo dell'immigrazione). Lo fa Presidente, e lo facciamo, in un tempo, come dimostra anche l'inizio di questo dibattito e il dibattito di ieri alla Camera, in cui è più facile alimentare le paure e speculare sul disagio che vivono ancora troppi italiani. È più facile animare una campagna elettorale permanente piuttosto che fare la fatica di dare soluzioni a problemi complessi, sapendo che le riforme, a partire da quelle fatte in questi anni, incrinano certezze, intaccano privilegi e hanno bisogno di tempo per migliorare concretamente la vita della persone che sono in difficoltà, un tempo che spesso rischia di essere percepito sempre come troppo lungo, come inaccettabile.

come stiamo facendo, a governare stando a servizio del Paese e degli italiani. Quello che votiamo oggi non è, non vuole e non deve essere un Governo per tirare a campare: ci sono obiettivi chiari e credo si possano ancora lavori non ancora terminati in Parlamento, che sono avanzati nel rapporto tra Stato e Regioni: penso alla riforma sul gioco d'azzardo e alla riforma del codice antimafia. È un impegno grande quello che si sta assumendo, Presidente, e che si assume il suo Governo. Ma forse l'impegno più difficile che si è assunto nella sua introduzione nella sua presentazione è quello di porsi l'obiettivo di provare a far tornare in questo Paese e in queste Aule un dibattito civile che rispetti le istituzioni: serve alla nostra democrazia. Alimentare lo scontro permanente, accreditare l'idea che tutto non funzioni, che tutto è un imbroglio e che questo è un Paese senza speranza rischia di rafforzare una deriva anti-istituzionale che non è né di destra che non è né di destra né di sinistra, ma è disperata e produce discredito su tutti. Una politica che si fonda sulla delegittimazione dell'avversario, non sul confronto e la proposta, non è una buona politica. Io sono convinto, Presidente, che lei e il suo Governo lavorerete per provare a riportare il confronto sulle cose e sulle soluzioni. Auguri, Presidente, a lei e ai suoi Ministri. Noi ci siamo. MPL))*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, che amarezza vedere come la classe dirigente di uno dei partiti più suffragati si sia trascinata in una estenuante lotta per il potere durante l'arco dell'intera legislatura: Marini, Prodi, Bersani, Letta, Renzi stesso, questa è la dolorosa litania di coloro che sono stati sacrificati pensando che il potere nel partito valesse quanto o più del destino della Nazione. Già, la Nazione, signor Presidente, la grande assente nel risiko degli ultimi tre anni: banche, scuola, giovani, lavoro, integrazione e tasse, parole diventate figurine di strategie di comunicazione che nulla hanno concesso in termini di spazio alla realtà. Una realtà dolente, che chiede buon governo e a cui voi proponete giochi di palazzo, facendo finta di allontanare Verdini per poter garantire a Renzi la supremazia al congresso del Partito Democratico. La realtà, però, non è il congresso del PD. In tanti condividevamo un giudizio ad inizio legislatura, motivando la disponibilità ad una grande coalizione: troppo grandi sono i problemi e gli ostacoli sul cammino dell'Italia! Occorre uno sforzo comune per rimuoverli, ma la storia successiva, quella del Governo Renzi, ha confuso la crisi dello Stato col saccheggio delle sue risorse, la valorizzazione del merito con l'occupazione della cosa pubblica da parte dei propri accoliti, il varo delle riforme con la creazione di regole che garantiscono al banco di vincere sempre. Il popolo ha reagito, recandosi in massa alle urne come non faceva da tempo, ha difeso come ha potuto libertà e democrazia paradossalmente, ha rifiutato il populismo dell'antipolitica del Governo difendendo le istituzioni, il loro significato, il loro essere garanti e non padroni della vita della gente. E voi cosa fate? Chiudete gli occhi, vi tappate le orecchie, fate un Governo che prende in ostaggio le istituzioni e che usate per differire l'esito della vostra mattanza interna. Rimuovete cioè lo scoglio delle riforme, abolendo il Ministero di riferimento, come quelli che aboliscono il reato di furto perché incapaci di prendere i ladri. Vi preparate al voto con una stravagante spocchia nei confronti delle opposizioni, «se siete capaci, fate voi la legge elettorale», con la malcelata intenzione di sabotare questo processo in modo da imporre risibili rifiniture dell'Italicum, dopo la sentenza della Corte costituzionale. Volete insomma che ci si arrivi senza poter realmente condividere la legge elettorale, perché una legge condivisa vi esporrebbe ad una sconfitta certa. Non ha quindi più senso interloquire con questa maggioranza, se non per stigmatizzare la lenta agonia che avete dispensato alla Repubblica: più *deficit*, più debito, più *caos* nella pubblica amministrazione e nella scuola, più arbitrio nelle carriere universitarie, più incertezza del diritto e, ovviamente, più tasse, molte più tasse, miliardi in più, sia nel 2015 che nel 2016. Ancor più tempo perso è riflettere sugli angosciosi 1.000 giorni del Governo Renzi, segnato da una sgangherata rincorsa al consenso fatta dissestando i conti dello Stato, scrivendo norme puntualmente rivelatesi incostituzionali, giocando a "disintermediare": parola è quasi comica, se non fosse che ha celato il primo tentativo della storia, da parte della politica, di dividere la società civile, separando, come nel caso di Confindustria e Coldiretti, l'opinione dei vertici dal sentire della base. Intervenire oggi, in questa sede, ha senso quindi se si disegna con pazienza e forza una possibile alternativa e la si indica con umiltà alla nostra gente . Mi rivolgo allora alle forze politiche, che nel solco della storia recente del Paese ne hanno retto le sorti, in alternativa ad una sinistra che oggi appare esageratamente ripiegata sulle proprie lotte intestine. Noi, appunto, non dividiamoci. L'Italia ha bisogno di un fronte politicamente coeso, in cui ci sia spazio per tutti, che rilanci il senso stesso della sovranità popolare e del ruolo indispensabile della nostra Nazione nel contesto euromediterraneo. Impariamo dai nostri errori e da quelli dei nostri avversari: è il popolo che sceglie la propria guida. Stiamo vicini alla nostra gente, ai loro bisogni, mostriamoci solleciti e leali con le difficoltà della Nazione e scopriremo che la nostra unità e idee nuove e ben ponderate saranno più utili all'Italia ed all'Europa di qualsivoglia concorso di bellezza per la *leadership* di un perimetro politico, che potrà essere tanto più ampio quanto più noi saremo inclusivi. Ribadendo il nostro «no» alla fiducia, signor Presidente del Consiglio, faccio al primo Governo assunto con i *voucher* gli auguri di buon lavoro, certo che un altro *referendum*, quello sul *jobs act*, sarà la vostra definitiva presa di coscienza della realtà del Paese. Signor Presidente del Consiglio, ognuno ha le proprie idee, ma io penso che l'articolo 1 della Costituzione obblighi il Parlamento e tutti coloro i quali hanno un ruolo istituzionale a prendere atto che il *referendum* del 2006 e poi quello del 2016 hanno stabilito che il popolo italiano ama questa Costituzione,

Bisogna fare una legge elettorale che deve essere innanzi tutto aderente alla Costituzione - non si può sbagliare su questo - nonché rappresentativa e in grado di assicurare la governabilità.

I parlamentari avranno l'obbligo di essere concreti e decidere in tempi ragionevolmente brevi. Signor Presidente, lei ha confermato all'economia il ministro Padoan, una persona di qualità professionale e morale. Mi auguro che il ministro Padoan impari dai numerosi errori che ha fatto per migliorare l'azione del vostro Governo, al quale io negherò la fiducia, ma che spero faccia bene per il Paese. Sul piano delle banche, di errori ne sono stati fatti molti; ne sono testimonianza alcuni dati di fatto. meritano il risarcimento per la questione delle quattro banche lo hanno ricevuto solo attorno al 15 per la riforma delle popolari è stata dichiarata forse incostituzionale dal Consiglio di Stato, non da noi. L'articolo di Giavazzi sul «Corriere della Sera» di stamattina mi esime dal dilungarmi nello spiegare quanti e quali lacune l'operato del Governo abbia avuto nella questione delle banche.

Signor Presidente, il Governo ha l'obbligo di agire, ma anche di sentire il Parlamento e di consentirgli di esprimersi con serenità, senza fiducie messe troppo a caso. Vorrei poi raccomandare, se ci fossero interventi dello Stato nell'ambito di Montepaschi o altro, che si abbia cura di verificare che gli *advisor* non guadagnino troppi soldi

mettono in evidenza la giusta volontà di dare vita ad un Governo che non svolga solo la pur fondamentale funzione di accompagnare il Parlamento all'approvazione di una legge elettorale, che riteniamo debba essere armonica tra Camera e Senato, e debba offrire, diversamente dall'Italicum, un giusto equilibrio tra rappresentanza e governabilità. Lei ha sottolineato la volontà da dar vita ad un Governo che si assuma anche la responsabilità di dare risposta alle principali emergenze del Paese: dai recenti terremoti, senza peraltro dimenticare anche quelli meno recenti dell'Emilia e dell'Aquila (le cui conseguenze ancora perdurano, seppure, ovviamente, con minore drammaticità),

ma richiederà anche parole e politiche chiare sulla qualità del lavoro. Garantire qualità del lavoro significa innanzitutto arrestare l'uso indiscriminato dei *voucher* e di altre forme che costano poco, in termini economici e di garanzie, rispetto al lavoro a tempo indeterminato. forme di impiego a cui le imprese ricorrono come scappatoia rispetto ad un serio impegno nell'innovazione, ma che tolgono dignità ai lavoratori e confinano, specialmente le giovani generazioni, in carriere intermittenti, poco retribuite, con poca contribuzione

di cui, unico assieme alla Grecia in tutta l'Unione europea, il nostro Paese è ancora privo. Vanno invece superate la frammentarietà e temporaneità di interventi come i *bonus*, poco pensati, poco coordinati, che disperdono a pioggia, con dubbia efficacia e sicura iniquità, le scarse risorse disponibili per le politiche sociali. Sbloccare e rinforzare la delega sulla povertà, ma anche altre normative che la lunghissima campagna referendaria ha bloccato (mi riferisco ad esempio alla legge sullo *ius soli*), deve essere un impegno congiunto e prioritario del Governo assieme al Parlamento. Particolare attenzione mi aspetto dal suo Esecutivo sul sistema sanitario: un sistema universale che deve garantire a tutti il diritto alla salute. Per questo mi aspetto, signor Presidente, un'accelerazione nell'approvazione definitiva dei nuovi livelli essenziali di assistenza e un impegno del Governo a monitorarne l'attuazione su tutto il territorio nazionale, come è suo dovere secondo il dettato costituzionale. Non ho capito, signor Presidente, se lei abbia deciso a chi affidare le delega sulle pari opportunità; eppure, in un Paese in cui, come ricordiamo ogni settimana qui in Senato, ogni 2,2 giorni una donna viene uccisa dal suo compagno o dal suo ex, il tema merita, anzi richiede, tutta l'attenzione dell'Esecutivo a partire dalla piena e paziente attuazione del piano contro la violenza. L'obiettivo della crescita, di una crescita inclusiva, richiede non solo - come da lei già ricordato - intransigenza nel contrasto alla criminalità organizzata, ma anche un presidio costante contro la corruzione, il clientelismo e la difesa della legalità. Il tema dell'evasione fiscale, del contrasto al caporalato e ad ogni altra forma di lavoro nero, così intimamente collegati tra loro, non possono che essere al centro dell'azione del Governo a cui daremo la nostra fiducia. ultimo, ma non per importanza, chiediamo al suo Governo di cominciare a impostare vere e proprie politiche industriali, che non si affidino soltanto a incentivi fiscali, tanto deboli quanto lo è la domanda, ma siano in grado di affrontare le criticità del nostro sistema produttivo e di dare prospettive al nostro sviluppo economico.

Signor presidente, colleghi, signor presidente del consiglio Paolo Gentiloni Silveri, desidero esprimere l'apprezzamento dei socialisti per lo sforzo che sta compiendo e per le fatiche che attendono lei e il suo Governo. Esecutivi che piacciano al 100 per cento è difficile averne: i Governi sono come le camicie confezionate su misura sul momento, tendono a rispondere ad esigenze del tempo, ma a volte hanno qualche grinza. Tuttavia anche le grinze, se non posizionate in maniera sconveniente, possono avere e dare carattere. Apprezziamo le sue messe a punto rispetto al dibattito prevalentemente portato avanti fuori dalle Camere, in particolare da parte di quanti non hanno voce in capitolo in Parlamento, ma giocano, magari cambiando casacca, la partita dei gufi e dei cosiddetti Concordo con lei sulle sue messe a punto costituzionali. Dobbiamo tornare al rispetto della Costituzione scritta confermata dal*referendum* del 4 dicembre. Signor Presidente, quanto è accaduto in queste ultime settimane dimostra che si può uscire rapidamente da una crisi di Governo e che si può rapidamente approvare nelle due Camere leggi importanti come quella di bilancio, senza eliminare la doppia approvazione di Camera e Senato. In particolare, il Senato, dopo la conferma del *referendum*, oltre a essere un'istituzione millenaria, ha dimostrato di essere un ventenne in grado di fare rapidamente chilometri di corsa che, in altre epoche, sono state risolti nell'arco di giorni. La sua abilità a rimettere in campo *verve* e senso di responsabilità è evidente. Credo che dobbiamo fare in modo che lei possa lavorare e che il Parlamento possa lavorare. non so se per volontà di Dio, della cui esistenza personalmente ho qualche dubbio, ma di altri della cui esistenza ho grande evidenza, è meglio che si superi il cincischiamento di questi ultimi mesi in attesa del grande evento che avrebbe dovuto cambiare la stagione di questo nostro Paese. nostro Paese. Come Parlamento dovremmo occuparci di alcune questioni di cui si parla da tempo e che riguardano direttamente la nostra capacità di muoverci con chiarezza e rapidità. I provvedimenti partono dalla considerazione che le grandi riforme, a volte, sono piccole cose rispetto alla fatica, ma di grande significato. Per quanto riguarda la prospettiva di questa legislatura, resto fedele all'imperativo di conseguire il più possibile la razionalizzazione e modernizzazione del meccanismo decisionale all'interno dell'assetto costituzionale esistente, fermo restando l'auspicio che la revisione costituzionale sia affidata, se si ritiene utile procedere a cambiamenti, in una futura legislatura secondo il metodo condiviso e proporzionale dell'Assemblea costituente. Da ora fino a fine legislatura le garantiamo l'appoggio

che in passato veniva tralasciata mentre noi abbiamo presentato in epoca non sospetta una proposta che recuperasse l'esperienza degli anni Novanta e Duemila

Nella presente legislatura vi è la possibilità di procedere mediante riforme regolamentari - in questo senso mi rivolgo agli assenti che erano per il no perché alcune modifiche di sostanza si potevano anche fare attraverso i Regolamenti e adesso è l'ora di modificare queste regole le esigenze di immediata messa a punto del procedimento legislativo. Ecco perché, alla proposta di modificazione del Regolamento del Senato, già da noi avanzata con il Documento II, n. 19, per la salvaguardia delle esigenze di governabilità del Paese, abbiamo aggiunto questa mattina un ulteriore un ulteriore contributo al dibattito per conseguire sin da subito un regime a parlamentarismo razionalizzato. si introduce per via regolamentare l'istituto della sfiducia costruttiva salvaguardando i poteri del Capo dello Stato, ma nel contempo vincolando i senatori a confermare per iscritto il nome del candidato *Premier* su cui intenderebbero dare la fiducia, in modo da alleviare anche la fatica

Si snellisce il procedimento legislativo con la prevalenza, in via ordinaria, della sede redigente. Si valorizza la stanza di compensazione nella negoziazione sugli atti amministrativi generali tra Stato e autonomie locali, anche mediante partecipazioni miste ai lavori degli organi di emanazione dei relativi esecutivi: *in primis*, la Conferenza Stato-Regioni. Si consente l'effetto acceleratorio, che finora è stato garantito dall'apposizione della questione di fiducia, con un miglior regime di contingentamento dei tempi e con un regime di urgenza che attiene alla trattazione dei soli disegni di legge provenienti dall'altra Camera. Si delimita la possibilità che i Gruppi che i Gruppi siano strutture volatili che operano a copertura di fenomeni di trasformismo parlamentare. Si rimette la disciplina della struttura del rapporto tra risorse umane e logistiche e beni strumentali alla normativa esterna. Questo, signor Presidente, perché l'autonomia di queste Camere deve essere rispetto ai contenuti delle leggi e non ai procedimenti amministrativi interni, che devono essere sottoposti alle leggi dello Stato. Non c'è extraterritorialità per nessuno, neanche per queste Camere. Almeno, questo è il mio punto di vista. Al Consiglio di Presidenza potrà essere consentito di approvare discipline derogatorie di singoli aspetti e della disciplina generale del pubblico impiego, motivate caso per caso per esigenze strettamente funzionali all'attività parlamentare e pubblicate immediatamente, per consentirne per consentirne l'immediata attuazione. Al di là di qualsiasi autodichia, rigidamente esclusa, l'eventuale sindacato giurisdizionale è su iniziativa di chiunque abbia interesse. Come vede, signor Presidente, c'è un lavoro, non solo per il suo Governo, non solo per questo Parlamento sui provvedimenti che lei riterrà opportuno debbano essere approvati, ma anche per una iniziativa autonoma del Parlamento rispetto alle questioni che nel dibattito referendario sono state poste e per le quali il sì e il no non potevano avere avere una risposta definitiva e assoluta rispetto a una posizione piuttosto che ad un'altra. Il buon senso deve portare a raccogliere le posizioni positive dell'una e dell'altra parte. Così come ha fatto lei, signor Presidente del Consiglio, recuperando una presenza di Ministri, di autorevoli colleghi, che hanno ben lavorato nel periodo precedente e che possono continuare a fare bene il loro lavoro fino alla fine della legislatura o, come ha detto lei, rispettando la Costituzione, fino a quando la fiducia del Parlamento ci sarà. *(Applausi

ho letto con attenzione il testo depositato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri e vi ho trovato parole e obiettivi che condivido; anche e soprattutto uno stile

In questo contesto è da apprezzare la rapidità con cui ha agito il presidente Mattarella: una velocità che è stata sostanza e che ha dato quelle garanzie indispensabili che l'Europa e i mercati chiedevano, con l'approvazione lampo della legge di bilancio e con un nuovo Esecutivo. Molti sono stati gli obiettivi raggiunti dal Governo Renzi in questi anni, anche di riforme attuate, meno mediatiche, come quella sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il superamento del Patto di stabilità;

al più presto, come la riforma della pubblica amministrazione, del processo penale o i provvedimenti come quello sul cyberbullismo. Sarà un Governo che affronterà, per il tempo che resterà in carica (ovvero fino a quando avrà una maggioranza che lo sostiene), a pieno titolo i problemi del Paese. Condividiamo profondamente il primo obiettivo che si è posto: l'intervento nelle zone colpite dal terremoto. Mi permetto, però, di ricordare anche la recente alluvione in Piemonte e Liguria. I cittadini e i Comuni di queste Regioni attendono con urgenza almeno la dichiarazione dello stato di calamità naturale e poi i provvedimenti successivi. Più in generale gli enti locali attendono quei provvedimenti che ci sollecitavano a inserire nella seconda lettura della legge di bilancio che non è potuta avvenire in Senato. Un eventuale decreto per gli enti locali dovrebbe affrontare il tema delle Province, per le quali si era ormai quasi concluso l'*iter* di trasformazione in ente di area vasta, con il completamento della riallocazione del personale, ma che dopo il risultato referendario tornano a essere a pieno titolo livello istituzionale. Va affrontato inoltre al più presto il tema dei precari dei centri per l'impiego degli altri settori. Credo sia molto importante l'impegno assunto dal Governo sul piano sociale: la crisi economica degli ultimi anni ha colpito cittadini e famiglie. Le misure del governo Renzi stanno portando risultati, con importanti inversioni di tendenza del prodotto interno lordo e dei posti di lavoro, ma la popolazione percepisce ancora poco di questi risultati. Una povertà crescente e la mancanza di lavoro hanno portato a un odio verso le istituzioni percepite come casta. Il fondo per la povertà, istituito nel 2016 e aumentato nella legge di bilancio per il 2017, è strategico, ma sappiamo bene che la povertà si risolve con più sviluppo e lavoro. Per questo trovo molto positivo l'impegno del Governo per la realizzazione delle grandi opere, con il nuovo piano straordinario dell'industria 4.0 e con un nuovo slancio della *green economy*. Mi permetto però di ricordare che è importante incentivare e sbloccare gli investimenti degli enti locali, perché i piccoli investimenti sono facilmente appaltabili in tempi brevi e con una diffusione su tutto il territorio. Ho molto apprezzato la volontà di un impegno per il Mezzogiorno. Mi rivolgo ai miei amici che abitano al Sud e non vedono decollare questa bellissima terra. Vada, Presidente, in queste zone d'Italia, come nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, perché hanno bisogno di sentire la nostra vicinanza. In attesa della riforma elettorale e del percorso interno dei partiti verso le elezioni, sono certa che il Governo farà tutto quanto necessario per le urgenze, ma non solo; i nostri giovani non possono aspettare neanche pochi mesi. E concludo: buon intenso lavoro, Presidente, a lei e a tutto il Governo. Governare e costruire è difficile; più facile distruggere. Se saremo, voi del Governo e noi parlamentari, sobri nei comportamenti, rigorosi e capaci di farci carico dei bisogni della popolazione, soprattutto dei più deboli e in difficoltà, i cittadini rispetteranno noi e le istituzioni che in questo momento ci è dato l'onore e l'onere di rappresentare. Infine, anche per me la passione è politica e, viceversa, la politica è passione. Sono certa che saprà, con la sua passione e la sua disponibilità, dialogare con i componenti della maggioranza, ma anche con quelli dell'opposizione, per il bene dell'Italia, delle donne e degli uomini del nostro Paese, soprattutto dei più giovani e dei nostri figli. Noi la sosterremo lealmente e con fiducia. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signora Ministro, colleghi, dato il ristretto tempo concessomi non mi dilungherò sui massimi sistemi e le porrò alcune questioni, rispetto alle quali sarà gradita una sua risposta nella replica, ma soprattutto nella sua attività di Presidente del Consiglio. i debiti della pubblica amministrazione: quasi tre anni fa il Presidente del Consiglio precedente promise il loro pagamento entro il suo onomastico del 2014, cioè il 21 settembre.

per il suo onomastico, signor Presidente, il 29 giugno prossimo, farà quello che non ha fatto il suo predecessore per i suoi tre onomastici precedenti? tre settimane fa il Piemonte è stato colpito da una grave alluvione, fortunatamente con pochissimi danni

calamità. Spero che la prossima sia quella buona; tutta la popolazione lo attende e anche l'intervento che mi ha preceduto ha richiamato questo punto. Terzo punto. Un Ministero che ha visto un importante cambiamento al suo vertice è quello dell'istruzione. Al nuovo ministro Valeria Fedeli va il nostro saluto, in quanto è stata fino a ieri la nostra Vice Presidente, e le auguro pertanto buon lavoro anche

per l'eliminazione obbligatoria dai libri scolastici dei cosiddetti stereotipi di genere? E tra questi stereotipi c'è lo stereotipo, che è

Sarà possibile avere una risposta su chi ha regalato dieci anni di concessione della Brescia-Padova, perché poi questa società privata se la rivendesse a una società straniera? Sarà possibile sapere come mai la Torino-Piacenza ancora non vede indetta la gara per il rinnovo della sua concessione, concessione, cosa che ci fa perdere almeno un milione al giorno, a danno dei contribuenti e degli automobilisti? Sarà possibile avere una risposta sulla Asti-Cuneo, che è una incompiuta peggiore della Salerno-Reggio Calabria? Infine, signor Presidente del Consiglio, nei confronti di Israele e dell'Iran: le due cose non possono essere disgiunte visto che l'Iran ha più volte promesso di distruggere lo Stato di Israele. Io conto sull'impegno da lei preso dopo lo sciagurato voto dato all'UNESCO negando l'importanza

islamico. Sul punto ci attendiamo che tenga fede all'impegno preso, anche se non capisco come mai nessun responsabile sia stato individuato. Dall'altra parte continuerà questa politica di incredibile apertura all'Iran, che ogni giorno (anche l'altro ieri attraverso il suo Ministro della difesa) ribadisce il suo proposito di distruggere lo Stato di Israele, ed ora, allargandosi abbastanza, anche gli Stati arabi del Golfo non sufficientemente schierati nel loro estremismo? Da tutte queste domande dipenderà evidentemente anche l'atteggiamento nei suoi confronti. In ogni caso, le auguro un buon lavoro nell'interesse degli italiani e del futuro del nostro Paese. Signor Presidente, presidente Gentiloni, le abbiamo già voluto dire ieri che abbiamo apprezzato i suoi toni più misurati, che speriamo possano essere davvero un punto finale rispetto all'arroganza e alla boria che purtroppo abbiamo dovuto sopportare in tutti questi mesi da parte del suo predecessore. Però le vorremmo anche dire con grande nettezza - ce lo consenta - che c'è davvero una distanza gigantesca, finanche siderale, tra questo tono più gentile e gli atti concreti di queste prime ore: la composizione del suo Governo, ma anche la sostanza delle cose che lei ha detto, che invece, a dispetto dei toni, sono in totale continuità con quello che è successo nei mesi passati e che purtroppo contengono ancora un elemento di fondo che davvero noi consideriamo difficile da comprendere, cioè una totale e assoluta rimozione di quello che è accaduto in questi mesi e di quello che è accaduto nelle urne di domenica 4 dicembre. Il vostro racconto è stato quello di chi non ha voluto vedere cosa stava accadendo nel Paese, quanto si allargasse in maniera sempre più clamorosa la faglia che pure da molti anni ormai attraversa la società del nostro Paese. Non solo, non avete voluto vedere che c'è un intero Paese, c'è un'intera generazione ormai completamente esclusa, tagliata fuori dalle scelte di fondo che la politica ha fatto per troppo tempo. nella composizione del Governo che avete voluto formare, il cosiddetto Governo fotocopia, e nei punti principali del programma che avete presentato davvero continuate a non voler vedere quello che sta accadendo. Eppure non ci voleva molto, presidente Gentiloni. ad esempio, osservare cosa è accaduto in tutti questi mesi quando il presidente del Consiglio Matteo Renzi visitava le varie città italiane: purtroppo per lui, invece di trovare il popolo a fargli scorta, così come raccontava, trovava manifestazioni, contestazioni, migliaia di persone che dal loro dal loro punto di vista tentavano di mettere in atto un elemento di profondo dissenso rispetto alle politiche del Governo. La verità è, Presidente, che avete operato una totale rottura con quel mondo che pure per decenni è stato il mondo della sinistra, dei progressisti di questo Paese. Avete rotto radicalmente con il mondo del lavoro perché avete voluto varare il *jobs act* e adesso tre milioni di lavoratori vi hanno ricordato, firmando la richiesta di un *referendum*, quanto profonda è stata la rottura con quel mondo. Avete rotto con il mondo della scuola: andate a leggere le percentuali relative ai flussi elettorali e vedrete quanti sono gli studenti universitari che hanno votato no al *referendum* costituzionale. Sono addirittura una percentuale ancora più alta di quella generale del Paese. Credo davvero che non basti semplicemente cambiare un Ministro a fronte del danno che purtroppo è stato prodotto. Avete rotto con quelli che per anni hanno tentato di difendere i territori in cui vivono, i comitati che hanno invano raccontato e detto in questi mesi che lo sblocca Italia ed il vostro comportamento irresponsabile sul *referendum* sulle trivelle erano anche quelli elemento di rottura con il Paese reale. poi rotto anche con quel mondo che pure esiste e che avete ancora una volta drammaticamente sottovalutato, anche dileggiandolo; quel mondo che per anni ha difeso la Costituzione di questo Paese, che ha respinto il tentativo di stravolgerla. Avete Avete anche inseguito la demagogia, facendo la cosa peggiore che si può fare in questi casi, perché se c'è una demagogia peggiore, presidente Gentiloni della demagogia dal basso, è la demagogia dall'alto, anche perché quando si utilizzano alcune parole poi inevitabilmente si fa la fine che avete fatto alle urne. Oggi con questo Governo fotocopia che avete voluto mettere in campo avete dimostrato di non aver proprio capito quello che sta accadendo nel Paese, né cosa sono quei 20 milioni di no, proprio come se quel voto non ci fosse mai stato. Non voglio neanche immaginare cosa sarebbe successo in Italia oggi se malauguratamente avesse vinto il sì, se nonostante i 20 milioni di voti fate finta di non capire quale disagio profondo cova in questo Paese, quanto la faglia si allarghi sempre di più e quanto un pezzo sempre più grande, soprattutto delle giovani generazioni, non si senta rappresentato da nessuno di noi. Eppure eravate stati voi a caricare quel voto referendario di un significato politico così grande e così forte, e allora sembra finanche surreale la composizione del Governo che ci avete presentato. Avete promosso i principali responsabili di questo disastro, quelli che davano persino il nome alla riforma. Ancora una volta avete agito in totale distonia con il sentimento del Paese, avete fatto il contrario di cercare di recuperare un elemento di connessione sentimentale che drammaticamente si è persa in questi anni. Signor Presidente, pur apprezzandoli - insisto - non bastano davvero i cambiamenti dei toni. Ci vorrebbe un cambiamento radicale della vostra narrazione. Ci vorrebbe un cambiamento radicale nel comprendere cosa è accaduto negli ultimi anni nei corpi sociali del nostro Paese. Questo vi ha detto il *referendum* della scorsa settimana.

proprio non si vede all'orizzonte, noi di Sinistra Italiana abbiamo detto fin dalle primissime ore successive al *referendum* quello che torniamo a dire adesso: naturalmente nessuna fiducia, anzi si faccia al più presto possibile la legge elettorale e si restituisca la parola ai cittadini, al popolo sovrano. E soprattutto lo si faccia con una legge elettorale che finalmente segni la parola fine rispetto alle leggi che ci sono state negli

perché la legge elettorale è problema di tutto il Parlamento, e non semplicemente della maggioranza di Governo. Mi pare di poter dire che il messaggio dei 19 milioni e mezzo di no su questo elemento sia molto chiaro: le regole non si fanno a maggioranza - ha detto quel voto

che con noi hanno depositato alcuni mesi fa il ricorso contro l'Italicum: è sbagliato pensare subito dopo il voto che quello che non andava bene ieri può andare bene oggi semplicemente per un interesse di bottega. Si metta una volta finalmente al primo posto e al primo punto il nostro Paese, che ne ha davvero bisogno. *(Applausi *(CoR)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio: finalmente. finalmente. Ci sono voluti più di due anni e mezzo per far capire alla classe politica che lo sosteneva l'inadeguatezza di Matteo Renzi a reggere quell'incarico che lei oggi rappresenta in Assemblea e per il quale si appresta a chiedere la fiducia. Vedere lei qui oggi, signor Presidente, è per me motivo di conforto, che mi deriva dalla consapevolezza che finalmente - uso un gergo popolare - la creanza ritorna sullo scranno più alto del Governo. Conosciamo il suo garbo, signor Presidente, la sua disponibilità al dialogo e al confronto, il rispetto per le ragioni degli altri. Mi creda, dopo anni di soprusi, forzature, angherie, di arroganza e maleducazione, tornare al normale confronto dialettico tra Governo e Parlamento è già un risultato. Fosse solo per questo, non esiterei ad accordarle la fiducia. Ma sappiamo bene che di questo non si tratta. Lei raccoglie, purtroppo, l'eredità di due anni di delirio istituzionale, due anni nei quali sono stati calpestati regole, regolamenti, diritti, rapporti, ragione e buonsenso. Questo è il raccapricciante dato della tanto osannata rottamazione renziana. E non si stupisca del clima che ci troviamo a vivere, signor Presidente. Ho avuto modo di ammonire quest'Assemblea - la cui ignavia ha permesso al dottor Renzi di maramaldeggiare tra e tra e nelle istituzioni - che, quando si calpestano i regolamenti, quando si mortificano gli spazi e i ruoli delle opposizioni, quando si irride alle ragioni degli altri, l'avversario politico diventa il nemico. E se l'avversario politico diventa il nemico, si è scavato un solco tale che riprendere il dialogo diventa impresa ardua. Apprezzo, quindi, il suo coraggio a raccogliere questa eredità. allora, che noi non ci aggiungeremo al coro di quanti sostengono che lei rappresenta il quarto Presidente non eletto; sarebbe come smentire noi stessi dopo la recente, affascinante e faticosa battaglia referendaria sulla Costituzione. Ma ciò premesso, abbiamo ben presente che gli italiani, oltre che la salvaguardia della Costituzione, hanno impresso con forza nel loro voto un messaggio di sfiducia nel Governo se posso aggiungere un'ulteriore considerazione sottovoce - anche un senso di sfiducia generalizzato, inviato un po' a tutti, affinché si ripristini un maggiore senso di responsabilità. Ecco, signor Presidente, l'Italia vuole una classe politica responsabile. Per fare questo, allora, bisogna recuperare serietà e verità. E, per recuperare serietà e verità, serve dare l'esempio. Signor Presidente, qui abbiamo iniziato male, allora. Indicare come Ministro degli affari esteri l'onorevole Alfano non è certo esempio di serietà, a meno che la gestione del caso Shalabayeva e dei molti altri casi che hanno costellato il mandato al Ministero dell'interno di due anni e mezzo siano motivo di giubilo, anziché di reprimenda. vedere giurare la senatrice Finocchiaro sulla Costituzione, nell'adempimento della sua nomina a Ministro, non è un grande esempio di verità. Io l'ho vissuta quasi come la peggiore blasfemia istituzionale. Questi sono due piccoli esempi di forma. dell'incarico al nuovo sottosegretario Boschi: taccio, avendo avuto la stessa molta più cronaca di quanta la sua mediocre storia meritasse. Nella sostanza, signor Presidente, lei ci rappresenta oggi le vere emergenze del Paese, che sono l'economia, il lavoro, il Sud - finalmente il Sud - e l'immigrazione. Queste urgenze, dimenticate nei due anni e mezzo precedenti, si sono purtroppo tramutate in emergenza. E, anche se noi le riconosciamo come obiettivo prioritario la nuova legge elettorale, sappia che se lei sarà capace di ristabilire il corretto e rispettoso rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento (se cioè eviterà di esautorare la nostra funzione legislativa e di indirizzo, inondandoci di decreti-legge) e se chiamerà la maggioranza che la sostiene a un maggior rispetto per le istanze delle opposizioni noi saremo disponibili al nostro contributo di idee e di confronto, rimanendo comunque fermo il nostro ruolo di opposizione.

del disegno di legge n. 1680, "Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università", con uno stanziamento - udite, udite - di 200 milioni di euro.

rendere obbligatori «i piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado» - quindi si comincia dalle scuole materne - adottando «misure educative volte alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza». Cito, ad esempio, l'istinto materno, che naturalmente non esiste ed è una sovrastruttura della politica. Quindi, fin da bambini bisogna educarli all'eliminazione di siffatti stereotipi. Naturalmente la sua nomina ha suscitato grande preoccupazione nelle famiglie, ma anche gli entusiastici applausi del circolo «Mario Mieli». E dico per l'ennesima volta in quest'Aula che il circolo «Mario Mieli» è intitolato a un noto sostenitore della pedofilia, a un cantore della pedofilia. pedofilia. Inutilmente abbiamo chiesto che il Governo Renzi interrompesse i rapporti con questo circolo, intestato a un noto pedofilo: speriamo che il nuovo Governo si decida a farlo. Noi abbiamo più volte denunciato, carte alla mano, il tentativo di colonizzazione ideologica della scuola pubblica e abbiamo più volte affermato, assieme a milioni di italiani nelle piazze del *family day*: «Giù le mani dai bambini». E ripeto in Senato: «Giù le mani dai bambini». Mi rivolgo oggi, nell'Aula del Senato, al nuovo Ministro affinché accantoni, da Ministro, i suoi progetti di quando era senatore. In caso contrario, è evidente che la nostra protesta e la nostra iniziativa politica saranno durissime in Parlamento e anche nel Paese. E credo che, dopo quello che è successo al *referendum*, che ha visto a quello che con sicumera e arroganza era stato sostenuto in questa sede, sfidando tutti a confrontarsi con il Paese, anche le certezze sulle sorti progressive - mi rivolgo anche al ministro Costa

Per quanto mi riguarda, è evidente che questo è un motivo in più per votare la sfiducia a questo Governo, nel quale devo dire, senza far nomi perché è sempre antipatico, troppi Ministri e Sottosegretari,

al *referendum*, si sarebbero responsabilmente ritirati a vita privata. E adesso, invece, li troviamo nuovamente seduti ai banchi del Governo. Signor Presidente, presidente Gentiloni Silveri, onorevoli colleghi, è opportuno ricordare a tutti, e anche a coloro che hanno sostenuto fuori e dentro il Parlamento altre tesi, che siamo in una Repubblica parlamentare e che i Governi si formano con i voti di fiducia ottenuti in Parlamento e durano finché la mantengono. Questo concetto e principio esce rafforzato dal risultato referendario che ha, per certi versi, fortemente arginato le spinte ipermaggioritarie e di modifica dei rapporti tra Governo e Parlamento. Vogliamo smentire quanti tra le forze politiche e sociali rappresentative del nostro Paese dichiarano demagogicamente che il nuovo Governo sia illegittimo in quanto non eletto dai cittadini. Il presidente Mattarella ha operato con sagacia e perizia, e soprattutto nel pieno rispetto delle regole costituzionali e delle prerogative proprie della sua funzione, avviando il giusto percorso indicato dalla nostra Costituzione, superando in tempi celeri una crisi che non ci avrebbe consentito di continuare a lavorare ai temi urgenti, politici, sociali ed economici e onorare gli appuntamenti sovranazionali in programma, risolvendo così con alto senso di responsabilità, in un momento difficile del nostro Paese, una delle più brevi crisi di Governo della storia della nostra Repubblica. La richiesta di andare subito al voto è insensata, inconcepibile e dannosa per il nostro Paese, poiché per assicurare la governabilità della prossima legislatura è necessario lavorare in Parlamento per arrivare, con il concorso di tutti i Gruppi parlamentari, a una legge elettorale che armonizzi i due sistemi di Camera e Senato. inoltre necessario che il nuovo Governo affronti le altre urgenze evidenziate dal presidente Mattarella, che riguardano i temi sociali ed economici e gli impegni europei e internazionali. Lo stesso presidente Gentiloni Silveri, nelle dichiarazioni programmatiche al Parlamento, ha rimarcato l'urgenza di dare all'Italia un Governo nella pienezza dei poteri, per rassicurare i cittadini e affrontare con massimo impegno e determinazione le priorità internazionali, economiche, sociali, a iniziare dalla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. La nostra condivisione al percorso seguito dal Presidente della Repubblica e alle sue scelte, il sostegno al governo Gentiloni Silveri, è frutto di tali valutazioni, ovvero di mettere subito mano ai «lavori in corso» del Paese, continuando a lavorare e rispettando impegni e scadenze programmati e indifferibili, senza sprecare il lavoro svolto dal Governo passato e senza perdere altro tempo. *Tempus edax rerum* dicevano i Romani: il tempo divora ogni cosa, ed è questo il rischio che non si poteva correre, che non possiamo correre e che noi non vogliamo correre. Il nuovo Governo si trova un Paese, una società e un'economia spaccata, caratterizzati da diseguaglianze rapidamente crescenti e da una ripresa ancora troppo debole. Si tratta dei divari tra redditi alti e bassi, tra generazioni giovani e generazioni anziane, tra settori produttivi e aree geografiche. Il nuovo Esecutivo dovrà indicare una strada seria trovando soluzioni e ricette a questa grande questione sociale: un italiano su quattro sfiora la soglia della povertà e nel Mezzogiorno il dato è ancora più grave. Si tratta di elementi che mettono a rischio la coesione sociale, provocando rotture e divisioni in profondità al nostro Paese. È il segno di una società che sta perdendo i suoi legami nazionali e generazionali, in particolare i giovani e tutto il Sud che si sentono abbandonati. Questa parte del Paese, anche attraverso il *referendum*, ha gridato a gran voce che non ce la fa e non vede luce oltre il buio del presente. Il nuovo Governo non potrà sottrarsi alla necessità di dare da subito una risposta efficace, concreta, tangibile a questo grande malessere. La crisi sociale è più grave della crisi economica. Uscire dalla recessione non vuol dire che la crisi sia finita. La crisi ha provocato un incremento del numero delle Servono politiche di vario tipo per affrontare questa emergenza, politiche attive del lavoro, di sostegno al costo dei figli e strumenti specifici di lotta alla povertà. La prima sfida di questo Governo - e credo che la costituzione del Ministero per la coesione e lo sviluppo del Mezzogiorno abbia questo fine primario dovrà essere quella di ridurre in maniera consistente le diseguaglianze ed evitare che la persistenza della povertà cresca e si consolidi. Signor Presidente, cari colleghi, il nuovo Governo, però, dovrà innanzitutto lavorare all'emergenza terremoto terremoto e il Parlamento alla nuova legge elettorale. Quella del terremoto è una chiara priorità che non può avere colore politico né subire logiche di palazzo. Dopo il terremoto del Centro Italia sono infatti oltre 16.000 le persone assistite dalla Protezione civile in sistemazioni provvisorie, persone che hanno urgenza di avere un alloggio stabile. Trovandoci ancora in piena emergenza, una lunga crisi politica non avrebbe certo giovato alle popolazioni del Centro Italia, che invece necessitano urgenti interventi da parte del Governo che possono arrivare soltanto con la stabilità politica. Arriviamo ora all'altro tema che rappresenta una priorità: la riforma della legge elettorale. Siamo di fronte alla più urgente scadenza politica nell'agenda del Parlamento. Attualmente abbiamo due sistemi diversi, uno per la Camera (l'Italicum) e uno per il Senato (il Consultellum). Il 24 gennaio la Consulta dovrà esprimersi sulla costituzionalità dell'Italicum. In caso di possibile e forse anche di probabile bocciatura di alcune sue parti, il Parlamento dovrà lavorare per avere una legge elettorale. Appare quindi irresponsabile la posizione di alcune forze politiche che chiedono di andare subito a nuove elezioni con le leggi elettorali vigenti perché - come ci ricorda il costituzionalista Ainis - avremmo un sistema schizofrenico con esiti opposti nelle due Camere legislative, che determinerebbe il "carnevale della democrazia". Altro impegno prioritario del nuovo Esecutivo sarà quello di sviluppare una politica a sostegno del sistema bancario. Il nuovo Governo dovrà affrontare la patata bollente dell'eventuale ruolo pubblico nel salvataggio del Monte Paschi, che non avrebbe certo conseguenze leggere sul bilancio dello Stato. Il problema del Monte Paschi va subito affrontato poiché, tra l'altro, si rischia un effetto domino tra i vari istituti di credito nazionali. E pur essendo il sistema bancario italiano sostanzialmente solido, tale solidità dovrà essere salvaguardata con linee guida per interventi successivi che si sperano non necessari. Infine, il nuovo Governo trova in agenda importanti appuntamenti d'ordine politico ed economico sia in Europa che a livello internazionale. Già domani si riunirà a Bruxelles il Consiglio d'Europa, l'ultimo del 2016. Al centro dei colloqui ci sarà il problema gravissimo dei migranti, che è stato lasciato tutto sulle spalle dell'Italia, e in particolare le nuove norme sul diritto d'asilo. Si tratta di un appuntamento fondamentale per l'Italia per richiamare l'Europa agli impegni presi sulla redistribuzione dei migranti. Altro importante appuntamento sarà quello che il prossimo 20 marzo vedrà a Roma le celebrazioni europee del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma. Infine, da gennaio per dodici mesi l'Italia avrà la Presidenza del G7, la cui riunione più importante si svolgerà tra il 26 e il 27 maggio del 2017 in Italia a Taormina, un evento che porrà il nostro Paese al centro della ribalta mondiale e potrà influenzare il nostro assetto economico. Appare superfluo ricordare che, a tali appuntamenti, l'Italia deve essere pronta e con un Governo ben definito, legittimato e che operi nel pieno delle sue funzioni. Detto ciò, signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo questo mio intervento anche a nome del Gruppo Area Popolare dichiarando che, coerentemente con quella che è stata la posizione assunta in questa legislatura di assicurare la governabilità al Paese e dando ancora una volta prova di responsabilità, esprimeremo la fiducia al nuovo Governo guidato dal presidente Paolo Gentiloni Silveri.

dalla poca discontinuità con il Governo precedente in merito alle sostituzioni e agli spostamenti. Credo che occorra fare un passo avanti nella valutazione di tutto questo, perché in questo momento deve essere protagonista la responsabilità politica, la responsabilità politica, che richiede uno sguardo concentrato sui contenuti e lucido sulle prospettive. Il suo tratto umano, prima ancora che politico, e la sua storia personale, signor possano offrire un profilo di affidabilità e garanzia per le sfide internazionali e le problematiche e le emergenze urgenti interne al Paese. Non è il momento degli effetti speciali e degli *slogan* e non è neanche il momento dei banchi vuoti: è il momento della partecipazione. La propaganda a lungo andare stanca e diventa noiosa. Spero invece che il Governo, dato per provvisorio e a scadenza - ma sappiamo che tutte le cose provvisorie durano più del previsto

da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale». È stato un grave errore dimenticare che esistono materie costituzionalmente tutelate da una riserva di Assemblea, come nel caso della legge elettorale, approvata solo perché il Governo ha posto più volte la fiducia. Ma i nodi prima o poi arrivano Occorrono governabilità e responsabilità. Quando la Corte costituzionale non sana le violazioni costituzionali, allora è il voto popolare che pone la sanatoria, come è avvenuto nell'ultimo *referendum*, allorquando il popolo italiano ha

malato che non si è curato quando era tempo e a cui non si è impedito di ammalarsi. Faccio un esempio concreto: se ad ogni seduta di quei consigli provinciali - mi riferisco al Montepaschi - si dà un gettone di presenza di 800-1.000 euro, poi

quindi, paghi pegno e la banca ritorni al suo servizio. Da questo punto di vista ristrutturare significa anche operare una svolta, con una separazione del potere politico

in risposta ai tanti sbarramenti, ai tanti muri che impediscono alla dialettica parlamentare di sviluppare e approfondire i discorsi in modo

dove le istanze di tutti devono essere rappresentate. Spero che questa sia soprattutto la sintesi della volontà dei cittadini che noi tutti, in modi diversi, e con Gruppi diversi, qui rappresentiamo.

questa è una legislatura difficile, politicamente complicata, dove momenti alti di responsabilità istituzionale si sono, purtroppo, miscelati con i più censurabili egoismi di personale politico vecchio e nuovo. Noi abbiamo rispetto per il nostro popolo. Abbiamo difeso in quest'Aula e nel Paese la sua sovranità. Per questo non accettiamo e non accetteremo mai pratiche di destrutturazione del nostro sistema democratico e costituzionale, né palesi né mascherate. Abbiamo scelto da sempre come terreno della nostra iniziativa politica l'area democratica e progressista. In questo senso, facciamo nostra la preoccupazione del Capo dello Stato perché il Parlamento operi prioritariamente per la messa in sicurezza del Paese e delle nostre comunità. Troppe sono le sofferenze inascoltate, le difficoltà di vita delle persone nei territori interni, nel nostro Mezzogiorno e nelle isole. Da questo disagio diffuso si alimentano movimenti qualunquisti, pericolose pratiche nostalgiche, veri rischi per la democrazia, per il bene dei lavoratori e delle loro famiglie. Noi siamo gente che ha radici, che rappresenta donne e uomini veri, in carne e ossa; non siamo un'immagine televisiva né una casualità telematica. Per questo contrastiamo con forza l'idea che mira a stravolgere i valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della partecipazione e dell'autonomia che sono sanciti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della Costituzione. Presidente, avremmo potuto lucrare sulle posizioni politiche legittimamente sostenute in questi anni di opposizione, accomodarci tra coloro che gridano vittoria e rispondere no alla chiamata di responsabilità e di condivisione. E, invece, stiamo valutando, riflettendo sul valore del nostro voto, che sarebbe contro corrente e non conformista. Stiamo valutando su quanto esso potrebbe tradursi nell'innesco della necessaria rivitalizzazione del campo progressista, interpretato non come uno sterile prolungamento della storia della sinistra italiana, ma come uno spazio partecipato per la costruzione di un futuro sicuro, di migliori condizioni di vita, di più giustizia sociale.

in condizione di sicurezza democratica, chiediamo un impegno vero, concreto e misurabile a favore delle zone interne e del disagio, del Mezzogiorno, della disoccupazione acuta e del diritto al riscatto nello sviluppo. particolare per la Sardegna, chiediamo il riconoscimento della loro condizione di insularità, la definizione di un nuovo regime di aiuti in linea con le disposizioni applicabili alle regioni europee ultraperiferiche. Chiediamo il riconoscimento dei medesimi diritti a tutte le minoranze, la ratifica della convenzione sulle lingue minoritarie, per una vera

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, credo che questo dibattito sia principalmente rivolto alle forze politiche più che a un Governo che è nel solco del precedente, sul quale

La vostra nave spavaldamente guidata dall'ex Presidente è andata o non è andata a sbattere contro un *iceberg* dalle clamorose proporzioni soprattutto, contrariamente alle condizioni climatiche, era molto più consistente al Sud che al Nord del Paese? Ve ne siete resi conto o - come è successo in passato, quando una grande nave è andata a sbattere contro l'*iceberg* - continuate a suonare la stessa musica, non capendo che la vostra nave affonda? L'avete buttata in musica, è vero: il Presidente del Consiglio uscente si è riferito ai mille giorni di Baglioni, il Presidente entrante a «Se stasera sono qui» di Tenco e voi alla musichetta del Titanic che affonda mentre continuate a strimpellare non rendervi conto di quello che vi è capitato. Nelle scarne dichiarazioni programmatiche del nuovo Presidente è scomparso completamente il tema delle tasse, della diminuzione della pressione fiscale,

Scompare il tema delle riforme, quando forse bisognava prendere atto dell'assoluta negatività della riforma costituzionale immaginata da questa maggioranza. Io, infatti, non voglio credere a chi butta tutte le colpe addosso al Governo, pensando di potersi lavare la coscienza dai banchi dell'opposizione. Voi avete votato

È scomparso il tema delle riforme quando si potrebbe riprendere immediatamente, perché vorremmo che si facciano attraverso una legge costituzionale che, alla prossima tornata, consenta agli italiani di eleggere una nuova Assemblea costituente assieme al nuovo Parlamento, sanzionando così definitivamente il fatto che i Parlamenti, soprattutto con premi di maggioranza, non sono adatti a fare a fare ampie riforme della Costituzione. Occorre, invece, un'Assemblea a se stante, che sappia ragionare in termini di rappresentanza proporzionale e assoluta di tutte le esperienze e le sensibilità politiche del Paese.

E se leggessero i *social* anche gli amici del Nuovo Centrodestra, si renderebbero conto di come stanno oltrepassando definitivamente un guado: transitano da una destra che non è giusto compaia più nel loro simbolo

per dire che non siete integrati nella sinistra del Paese. Prima c'è stato il Governo Monti con le larghe intese condivise;

le riforme. Adesso che gli italiani hanno bocciato la riforma mi chiedo qual è la scusa che avete per non dichiararvi direttamente organici al centrosinistra. Il discrimine forte che gli italiani vedono politicamente in questo cambio di Governo, per quanto ci riguarda, sta proprio nel vostro definitivo passaggio al centrosinistra. Alle prossime elezioni non potete pensare che si

l'espressione chiara che la stabilità dei Governi dipende non dalle leggi elettorali, ma dalla coscienza dei singoli parlamentari fin quando esisterà, come esisterà anche per la prossima legislatura,

al nuovo Governo, risiedono nella coscienza dei singoli parlamentari e, purtroppo, sono svincolati dalla volontà popolare. Una cosa è certa: la volontà popolare in questi giorni è chiara e netta. Si è espressa soprattutto al Sud del Paese

ampi strati sociali del Paese, ampi territori del Paese e che ha condannato - come il senatore Uras ha fatto riferimento alla Sardegna, consentitemi di fare un brevissimo accenno alla mia Sicilia mia Sicilia - la Sicilia a un Governo che la sta distruggendo definitivamente. Ancor di più, il combinato disposto tra Governo regionale e nazionale sta definitivamente cancellando la speranza di un vero progresso e sviluppo economico. anche su questo. Rifletta soprattutto la maggioranza che la sostiene: continuare a sostenere un Governo come quello che per ora sta amministrando la Sicilia, significa voler far male ai siciliani e, politicamente, far male a voi stessi e ve ne siete resi conto - spero - con il risultato referendario.

un Governo con un Parlamento; deve riconciliare un Governo, e insieme il Parlamento, con il Paese. di rotture, ad anni di imposizioni, ad anni di stravolgimento di regolamenti, anche parlamentari, a forzature e a *spot*, uno dietro l'altro. Qualcosa di incredibile, che dovrebbe portare tutti a ragionare e a dire che le forzature avvenute in questi anni non devono diventare la regola nella prossima legislatura. La coscienza di ognuno di noi, di maggioranza e di opposizione, dovrebbe condurre a riportare sul serio il Parlamento al centro di tutto inizia con il rispetto da parte di un Presidente del Consiglio, che è qui, che ogni tanto ci guarda e ascolta anche l'ultimo di noi, che semmai sono io, e che, semmai, dice qualcosa in una eventuale replica. Questo non è mai avvenuto: c'è chi veniva qui,

E ha fatto poi riforme assurde. Riforme fatte per farle, come quella delle Province e vorrei dire al ministro Delrio, che è qui, che sarebbe ora che bloccasse i procedimenti di votazione ancora in corso. Bisogna ragionare. Si ritorni un po' indietro, perché anche quella della Province è un'altra riforma *spot*,

vivere un'esperienza parlamentare di Governo dicendo sempre no a metà del Paese su qualsiasi argomento, non disposti recepire mai nulla? Questo è il compito principale che lei ha

Lo dico con serenità, perché quello è un segno di rispetto, non verso di me, ma verso quest'Aula e quello che vuol dire ed è su questo che noi la giudicheremo, perché è tutto da rifare. Detto con serenità: noi voteremo contro questa fiducia. siamo usciti fuori da una forza politica a causa della riforma costituzionale e dell'Italicum, a mani nude. Non abbiamo contrattato nulla con nessuno, per una coerenza e una dignità che appartengono al ruolo di un parlamentare. Questo è il dato reale.

spetta alla sua serietà, spetta a quel che farete e proporrete, se tutto questo viene recuperato. Fino ad allora staremo qui a stimolare, a fare l'opposizione che ci compete, in termini duri, politici, ma mai offensivi verso nessuno, pronti a sostenere le cose giuste, che finora non abbiamo visto: su tutti gli argomenti siamo disposti a ragionare. Poi sinceramente, Presidente, alcune figure che ci sono nel Governo ve le potevate risparmiare. Sono figure che sono state arroganti tanto quanto l'ex Presidente del Consiglio e ora stanno qui. Mi auguro che non abbiano compiti molto delicati. Lo dico qui: stiamo attenti a chi diamo

come si dovrebbe fare nel momento in cui si inizia, ci sarebbe da leggere l'appello, con i presenti e gli assenti. Spiace certamente che oggi non sia presente la senatrice Finocchiaro, neo ministro delle riforme e dei rapporti con il Parlamento, anche per il ruolo stesso che ella ha deciso di rivestire in questo Governo; spiace che non ci sia più il ministro Costa, che non ci sia il ministro dello sport Lotti, che evidentemente è impegnato fuori a contrattare i posti da Sottosegretario. Spiace che non si sia neanche fatto vedere il ministro degli affari esteri Alfano. Il ministro degli affari esteri Alfano: sì, perché dopo avere devastato l'interno, adesso ce lo troviamo anche agli esteri. Spiace che non ci sia il ministro della giustizia Orlando; spiace che non abbia neanche messo piede in Aula questa mattina il ministro Padoan, per non parlare del ministro dello sviluppo economico Calenda. È venuto fugacemente e se ne è subito andato il ministro Martina, neanche è entrato in Aula il ministro Galletti, il ministro Delrio è entrato e uscito, il ministro del lavoro Poletti è non pervenuto, il Ministro dei beni culturali è arrivato poco fa, ma adesso è già scomparso. E certamente manca la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Elena Boschi.

Voi oggi rappresentate essenzialmente una fotocopia del Governo Renzi: un Governo che, come abbondantemente noto, è stato costruito nelle segrete stanze del Nazareno,

Vede, Presidente, lei avrebbe avuto la possibilità di dimostrare, anche per la sua storia e la sua personalità, una discontinuità. Le riconosco una differenza: almeno, rispetto al suo predecessore, non prende il caffè in Aula, ma l'attenzione che meriterebbe qualsiasi intervento che si svolge qui in Aula vedo che continua a mancare.

dall'esito del *referendum* è quella dei 20 milioni di cittadini che hanno detto no. Hanno detto di no all'arroganza del presidente del Consiglio dei ministri Renzi, ma hanno detto no in maniera esplicita alle politiche del Governo Renzi, alla compagine dei Ministri che ha costituito quel Governo e che ha condotto gli italiani a perdere fiducia e a dire no in maniera secca a politiche che hanno illuso sul lavoro, creando invece sudditanza dei lavoratori con i *voucher*, a politiche che hanno illuso sulla scuola creando semplicemente una grande confusione, a politiche che avrebbero avuto la pretesa di riformare la pubblica amministrazione, producendo, in effetti, solamente forse una pagina - dico male, senatore Calderoli? - perché, forse, solo il codice digitale è rimasto vivo di quella riforma, visto che è stata dichiarata incostituzionale. Sotto la scure della Corte costituzionale c'è anche la cosiddetta riforma delle banche popolari, perché quando avete messo mano al sistema bancario, lo avete fatto per tutelare gli amici e i finanziatori o lo avete fatto per disfare, là dove funzionava, il credito ai piccoli risparmiatori. Oggi la Corte costituzionale giudicherà il vostro lavoro e anche questa volta, purtroppo, sappiamo di aver perso un'ennesima occasione di serietà. L'avete persa. Chiedo a lei dov'è la serietà, nell'andare a nominare come ministro degli affari esteri Alfano, un ministro che all'estero non so come possa rappresentare degnamente un Paese che non ha saputo difendere all'interno. Ecco il ministro Alfano che arriva, è arrivato al momento giusto. Ministro Alfano, si accomodi, ce n'è anche per lei, non stia in pena. E magari prenda qualche lezione di inglese, perché l'ultima volta che ha dato qualche esempio, non è andato sulle cronache con gli applausi, ma con molta ironia, purtroppo. Noi ci aspettiamo un Governo che invece vada a difendere gli interessi del Paese in Europa, che non sia piegato rispetto agli interessi della Germania, che non sia piegato rispetto agli interessi che sul nostro Paese si sfogano, come vediamo in queste ore, utilizzando il sistema finanziario come leva per acquisire e per entrare pesantemente nel nostro Paese. Voi avete fatto pagare un prezzo pesante, con le contraddizioni, le ipocrisie e le falsità di Renzi e quelle del Partito Democratico, un prezzo già troppo elevato fino a ieri, ma da oggi ancor più elevato. Abbiamo bisogno di elezioni. Non abbiamo bisogno di elezioni per uno sfizio, ma perché il Paese non può permettersi dieci, dodici o quindici mesi di campagna elettorale costante, sfibrante, con scelte fatte non in ragione delle necessità del Paese, ma in ragione delle tensioni che all'interno del PD si svilupperanno o dovranno essere gestite e diluite con gli alleati che vi troverete in questa o nell'altra Aula, a seconda delle convenienze. *(Applausi della senatrice Bignami)* Questo non è ciò di cui ha bisogno il Paese. Il Paese ha bisogno della stabilità di un Governo che sia finalmente espressione di una volontà popolare, che nasca finalmente da una maggioranza eletta dal popolo, non da una maggioranza comprata con gli strapuntini di Sottosegretario in Parlamento, perché questo sarebbe l'ennesimo schiaffo dato ai cittadini. Non sappiamo quanto durerà il Governo. Lei, presidente Gentiloni Silveri, ha Ci sono certamente degli inciampi sul percorso del Governo che credo segneranno in maniera mortale questo percorso e non mi riferisco all'interesse dei cittadini, che sarebbe quello di andare a votare domattina, ma al *referendum* sul *jobs act* e sui *voucher*, che vi aspetta alla prova di giugno. Quella sarà veramente una prova con la quale vi accorgerete nuovamente quanto il Paese è lontano rispetto a quello che avete descritto via *tweet* o con le *slide* a inizio legislatura. In questo Governo continuano a sedere Ministri di fedele credo renziano, che invece di affrontare i problemi del Paese hanno creduto che per governare bastasse illudere il popolo con false riforme, forti del consenso ruffiano di un *establishment* corporativo che rappresenta al massimo solo se stesso; un consenso cortigiano che abbiamo visto in occasione della campagna elettorale per il *referendum*, espresso e sostenuto da *opinion leader* come il presidente di Confindustria, quello della Coldiretti o di altri sindacati: esponenti di una dirigenza incapace di intraprendere e capire oggi i problemi del Paese reale, lontana dai problemi del lavoro ma attenta a cementare rapporti di potere personale. Questo è un Governo, come efficacemente notato ieri da Massimo Franco sul «Corriere della Sera», il cui livello di lealtà a Renzi è fin troppo dimostrato dalle riconferme dei Ministri: come è stato abbondantemente detto, una brutta fotocopia del precedente Esecutivo. Vorremmo avervi davanti, invece, come un Governo che si regge su una maggioranza legittimata dal voto popolare, un voto che avete tradito, come avete tradito nei mille giorni trascorsi a curare prima le *slide*, poi i *tweet* e poi la comunicazione con i comunicatori assunti da oltreoceano. I problemi di cui vorremmo parlare sono quelli di un Paese in cui il 40 per cento dei giovani resta disoccupato, in cui, Presidente, 100.000 giovani se ne sono andati lo scorso anno all'estero, sperando di trovare quel lavoro che il loro Paese nega loro in patria. Un Paese nel quale il Governo è parte attiva in un sistema devastante che, dietro la parola «accoglienza» procaccia affari con un fatturato di quattro miliardi, riempiendoci i paesi di immigrati clandestini che, quando va bene,

«Tutti i debiti della pubblica amministrazione» disse «o andrò in pellegrinaggio a piedi». Sappiamo che non ha mantenuto quell'impegno, come ben si è guardato dall'allontanarsi dalla politica come aveva più volte dichiarato se avesse perso il *referendum.* Lo stesso ha fatto la sua fidata Maria Elena Boschi, oggi nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da cui passeranno tutte le nomine negli enti partecipati dallo Stato nei prossimi mesi, da cui passeranno tutte le scelte fondamentali ed anche i *dossier* che riguardano le banche, e penso al grande scandalo di Monte dei Paschi, che avete tenuto da affrontare dopo il *referendum.* Questa è stata la logica che ha contraddistinto l'operato del Governo Renzi di cui ancora oggi lei si assume la responsabilità, confermando quelle persone in ruoli chiave: prendere gli italiani in giro. Non vi è bastato a comprendere che il risultato del *referendum* dice che la gente ha voglia di democrazia, ha voglia di scegliere, ha voglia di decidere. La gente è stufa di un Governo che gli dica: «Alle Province cambiamo nome, togliamo le elezioni, ci pensiamo poi noi politica a gestirle». La gente vuole scegliere, la gente lo ha detto respingendo la vostra riforma costituzionale. La gente non vuole norme di supremazia che dicono che il Governo decide per tutti. La gente vuole contare, il popolo vuole contare. Capite questa lezione e si vada velocemente al voto, ridando forza elettorale ai cittadini. Siano loro a decidere il programma del Governo, non siano gli interessi di chi siede sui banchi dei Ministri. Voi avete bypassato troppe volte il consenso elettorale, pensando di farvene gioco. Presidente, questo è un Paese lacerato, è un Paese che avete lacerato con la campagna elettorale, è un Paese che avete diviso classificando per buoni quelli che votavano sì e per cattivi quelli che votavano no, che avete definito gufi, retrogradi, poltronari, solo perché dall'altra parte c'era un arrogante Presidente del Consiglio dei Ministri. Nei pochi mesi che ci auguriamo duri questo Governo, faccia almeno questo sforzo: sia il contrario rispetto a Renzi, abbandoni quell'arroganza che ha contraddistinto il Governo Renzi, perché quell'arroganza è stata respinta da 20 milioni di cittadini. Nel suo richiedere di abbassare i toni, rivolga queste indicazioni innanzitutto al suo segretario politico, che ha - ripeto - diviso il Paese tra buoni e cattivi in un momento in cui, quando si parlava di Costituzione, sarebbe invece stato dovere di uno statista unire il Paese.

rispetto alla legge elettorale ed alla volontà di andare velocemente alle urne? Perché lo avete dimostrato in passato: la legge elettorale che oggi è in vigore, l'Italicum, l'avete costruita qui dentro e alla Camera con il manganello,

presidente Grasso: la sovranità appartiene al popolo! E lo grideremo forte in tutte le piazze, fino a quando le elezioni non saranno effettive. Voi continuate pure a trescare e a tramare alle spalle del popolo, pensando che nessuno se ne accorga; ma se ne accorge, eccome. Continuate pure a tutelare le *lobby* e quelli che vi finanziano. Noi, la Lega, resteremo invece nelle piazze, resteremo tra il popolo, resteremo nei paesi, grandi o piccoli, dove la gente vuole scegliere, dove la gente vuole decidere, dove la gente vuole contare, dove la democrazia ha già vinto dicendovi per 22 milioni di volte no.

consultazioni avviate dal Capo dello Stato: di fronte alla proposta, avanzata dal Partito Democratico, di formare un Governo allargato alle forze dell'opposizione, alle forze che avevano vinto il *referendum*, anche come segno evidente di presa d'atto di una sconfitta determinata dal *referendum*, la Lega, proprio la Lega che abbiamo ascoltato ora, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno risposto no: non sono stati disponibili, non hanno voluto lavorare, oggi, nell'interesse del Paese. Questo Governo, con la consapevolezza dell'esistente, è una manifestazione di responsabilità delle forze di maggioranza, del Presidente del Consiglio, di tutti i deputati e senatori che voteranno la fiducia, per onorare una giusta esigenza posta dal Capo dello Stato. Lo stesso presidente Paolo Gentiloni Silveri, ieri, nel dibattito alla Camera, ha citato il titolo di una bellissima canzone di Luigi Tenco. Ecco, se stasera è qui, se oggi, se stamani è qui, è perché con il *referendum*

Una sconfitta, che però è anche di quest'Assemblea, signor Presidente, dal momento che la riforma bocciata dai cittadini qui è stata approvata ben tre volte, qui è stata discussa, qui è stata modificata, qui è stata migliorata, a mio avviso. Consentitemi di spendere due parole sulla scelta di Matteo Renzi, una scelta non molto praticata in Italia e che rende onore alle sue parole e agli impegni assunti. Matteo Renzi oggi, a differenza di tutti noi, non percepisce alcuna indennità e ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo dagli elettori del centrosinistra prima e dai cittadini poi, il prima possibile. È una decisione che onora e riscatta la politica e che dovrebbe essere apprezzata al di là dei banchi di appartenenza. Ci sono luoghi, signor Presidente, molto vicini a questo, non distanti da qui, mi riferisco al Campidoglio, dove per dare le dimissioni ci sono volute settimane e mesi, conoscendo informazioni che ormai erano patrimonio dell'opinione pubblica. Qua invece, la sera stessa dell'esito elettorale si è deciso di mantenere ciò che si era detto. E allora eccoci qua a votare la fiducia a un nuovo Esecutivo che, come ha detto il presidente Gentiloni Silveri, nasce in continuità con il Governo precedente. Mi ha fatto piacere ascoltare la priorità enunciata ieri alla Camera e che si trova all'interno del documento programmatico, enunciata con forza, ripetendo tre volte la stessa parola: lavoro, lavoro, lavoro. Ho apprezzato l'intervento del presidente Gentiloni Silveri: il lavoro al centro dell'attività di Governo, sapendo che si può contare su provvedimenti all'interno della legge di bilancio, come Industria 4.0, che prevedono investimenti e un rilancio del sistema economico, sapendo che il lavoro si produce solo se si ricrea ricchezza e se si rimette in moto un sistema produttivo che possa permettere all'Italia di essere nuovamente competitiva. Certo, guardandomi intorno, sono stupefatto: mancano dall'Aula alcuni Gruppi, quei Gruppi che dicevano di difendere la Costituzione e che con la loro assenza, a mio modo di vedere, la offendono oggi. Troppe volte, anche nel passato più recente, quest'Aula si è trasformata in un'arena, in un luogo dove non si esprime più la rappresentanza del Paese, ma dove semplicemente si vuole fare chiasso, rumore. Condivido la premura espressa dal Presidente sulla necessità di accompagnare le forze politiche nella riforma elettorale. Le forze politiche, quelle stesse forze politiche che ci dicono che presto si deve andare a votare, che subito si deve andare a votare; quelle stesse forze politiche che si dichiarano indisponibili affinché tutti insieme si possa andare a votare; quelle forze politiche che non si vogliono sedere a un tavolo per lavorare affinché le regole del gioco siano concordate e rese applicabili da subito. Mi viene il dubbio sull'effettiva volontà di quelle forze politiche di fare ricorso al corpo elettorale, come sarebbe giusto fare

ci sono uomini che servono il Paese. Noi sappiamo di poter contare su di lei. MPL))*. Signor Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio, l'Italia si è confermata un grande Paese. Il voto del 4 dicembre ha dimostrato che vi è un popolo libero e dotato di buonsenso; quel popolo che nella storia repubblicana si è sempre mobilitato di fronte al rischio di strappi e salti nel buio. D'altro canto, il fatto che oggi si formi un Governo senza che delle temute catastrofi si sia avvertita nemmeno una lontana eco sconfessa le ipotesi ultimative paventate perfino da chi istituzionalmente avrebbe avuto il compito di smentirle. L'Italia, signor Presidente, è un Paese libero e forte. Tuttavia oggi è anche un Paese sofferente e sarebbe un imperdonabile errore sottovalutare questo suo stato. Tra i tanti problemi, tre emergenze strutturali si segnalano per la loro intrinseca pericolosità. La situazione del credito, innanzitutto, sulla quale si è perso troppo tempo inseguendo scenari privi di riscontro. Non è ancora chiaro per quale motivo sul Monte dei Paschi di Siena siano state rigettate *a priori* ipotesi concrete di apporto di capitale privato, senza nemmeno verificarle, mentre ci si avvia verso una nazionalizzazione che graverà ulteriormente sui conti dello Stato. Non è chiaro quale linea si intenda adottare sulle quattro banche tecnicamente fallite Non è chiaro se, dopo lo *stop* del Consiglio di Stato sulla riforma delle banche popolari, il Governo intenda mettere riparo ai propri errori, a suo tempo invano denunciati, per evitare il rischio di ulteriori focolai di crisi. Signor Presidente, tutto ciò non è chiaro mentre in questo ambito urge chiarezza, anche rispetto ai rapporti che in passato vi sono stati tra il potere bancario e il potere politico. Senza credito non si può nemmeno parlare di ripresa e noi non possiamo pagare questo prezzo per coprire malefatte e comportamenti di dubbia legalità. Non meno ci preoccupano, signor Presidente, i conti della previdenza. Solo pochi anni fa abbiamo affrontato un intervento legislativo che ha inciso nel corpo vivo della Nazione, creando ingiustizie che pesano come macigni sulla coesione della nostra società. Dobbiamo oggi essere certi che i conti siano a posto, che non vi siano buchi o omissioni nelle comunicazioni che impongano poi ulteriori interventi d'urgenza, il terzo nodo strutturale fuori controllo è l'immigrazione. Agitare una battaglia paraideologica tra falchi e colombe serve solo a coprire un impressionante vuoto di politica. Perché la verità è che in quest'ambito l'Italia ha smesso di avere una politica quando ha pensato di poter contare sulla permeabilità delle frontiere dei Paesi confinanti. Ora, non c'è dubbio che il problema abbia una portata europea e addirittura che l'Europa vivrà o morirà proprio su questa emergenza epocale. Questo però non può diventare un alibi, né può giustificare il fatto che nel vuoto di politica nazionale ad avvantaggiarsi del dramma siano coloro che finiscono con l'arricchirsi. È arrivato il tempo di darsi una visione e soprattutto una linea di intervento che sollevino le popolazioni dalla sensazione di essere esposte ad ogni tipo di imprevisto. Signor Presidente, queste emergenze strutturali indeboliscono ancor di più il tessuto connettivo del nostro Paese. Innanzitutto a livello sociale, laddove la crisi ha acuito le diseguaglianze e ha "spianato" il ceto medio, quell'operosa spina dorsale che ha sempre ricercato nel benessere proprio e dei propri figli un mezzo attraverso il quale accrescere il benessere comune. Sicché la stessa categoria del moderatismo ne ha risentito: oggi i moderati in questo Paese sono i più arrabbiati e chi ne rappresenta i sentimenti ha il dovere di comprenderne le ragioni, non per assecondarle acriticamente, ma per catalizzarle verso scelte costruttive. Il tessuto connettivo si è poi indebolito a livello politico, anche per l'illusione di poter risolvere la crisi inseguendo, dal palazzo, l'ondata dell'antipolitica. Sicché oggi sul piano dell'attacco alle istituzioni è difficile distinguere tra politica e antipolitica, con l'ulteriore conseguenza che quando ciò accade è sempre l'originale che vince sull'imitazione. Infine, la coesione è stata colpita a livello delle Istituzioni. Non sto qui a tediarla, Presidente, con il lungo catalogo delle forzature, delle illegalità, degli sbreghi messi in atto nel corso della campagna referendaria. Ma insistere su questo punto non significa infierire: significa ricordare affinché si possa mettere riparo. Questo è il punto, signor Presidente del Consiglio. Il suo Esecutivo sconta già in partenza il limite della sua composizione: uno schiaffo al voto degli italiani del 4 dicembre. Ora starà a lei decidere se assecondare fino in fondo l'ansia di riconquista del suo predecessore, piegando le scelte di Governo all'imminente campagna congressuale del PD, o rompere gli schemi, incaricandosi di avviare la ricucitura del tessuto di un Paese uscito lacerato da una vicenda lunga e sfibrante. L'atteggiamento da lei annunciato sulla legge elettorale è un buon segno ma, per l'appunto, è un segno. Serve ben altro. Presidente Gentiloni Silveri, l'ultima volta che ci siamo incontrati, prima del *referendum*, di fronte alle preoccupazioni per l'eccessiva personalizzazione della vicenda che la Nazione stava vivendo, lei mi disse di credere in una politica fatta da *leader* in grado di incarnare un messaggio e trasmetterlo alla Nazione, e auspicò che analogo schema possa tornare a prodursi anche nell'altro versante del sistema politico, al quale io appartengo. a tutto ciò credo anch'io, per antica fascinazione per il mondo anglosassone e le sue dinamiche e per la comprensione di quei fenomeni di modernizzazione che rendono il *leader* un necessario tramite tra le loro comunità di riferimento e la Nazione, sui quali per primo si esercitò Weber. Lei, però, oggi deve prendere atto che se è stato chiamato a guidare il Governo della Repubblica è perché quello schema al quale entrambi crediamo è fallito, non per la sua intrinseca debolezza ma per il modo con il quale, da ultimo, è stato interpretato: con insostenibile leggerezza, con ignoranza del portato storico di quel cambiamento, con inconsapevolezza degli obblighi istituzionali che lo devono sostenere. Si tratta ora di tornare pazientemente a riparare la tela oppure sfasciare definitivamente il telaio. Ognuno nel ruolo che si è scelto. Da oppositore al suo Governo, signor Presidente, le auguro di lavorare dalla parte dei ricostruttori. Non tanto per il bene dell'Esecutivo che lei guida, che non è in fondo un mio problema, ma per il bene del nostro comune Paese.

istituzionale, come atto di responsabilità verso il Paese. Alla stessa responsabilità il Parlamento dovrà fare ricorso per uscire dall'*impasse* in cui ci troviamo e mi riferisco, ovviamente, alla necessaria concordanza delle leggi elettorali.

che quelle parole rappresentano sia sentito come priorità strutturale di un Paese che, come lei dice, punta al lavoro, al lavoro, al lavoro. La crisi di Governo ha impedito che questo ramo del Parlamento affrontasse nel merito la legge di bilancio ed è rimasto così sospeso

che quell'impegno sia onorato dal suo Governo e che il suo Governo si intesti un atto di responsabilità verso l'intera comunità degli studiosi del nostro Paese, giovani e meno giovani, impegnati in campo umanistico e in campo scientifico, che confidano di avere l'opportunità di liberare le loro idee per il loro Paese e di metterle a disposizione. A quelle idee credo che dobbiamo doverosamente guardare per realizzare prospettive di sviluppo durature. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà. È una novità dopo tre anni nei quali il suo predecessore si presentava in queste Assemblee sfidandole, provocandole e chiedendo al Parlamento di obbedire ai *Diktat* dell'amministrazione, del Governo e delle *lobby* economiche che influivano sull'azione del Governo.

«la ricerca paziente, dal basso, di una politica meno arrogante, meno sicura di se, più «umile», anche più orientata alla ricerca dell'incontro al di là dello scontro, della convergenza possibile al di là della contrapposizione; più capace, anche per questo, di parlare il linguaggio della verità, magari scomoda, dell'unità e della solidarietà. Una politica che guardi avanti e in alto, pur mantenendo i piedi bene per terra e individuando i passi che si possono fare ogni giorno». Penso anch'io quello che scrive Onida, ma non ci siamo, perché il suo Governo contraddice i suoi toni garbati: è peggio di una fotocopia del Governo precedente. Ne fanno parte due signore, che peraltro apprezzo per le loro competenze, ma che hanno scritto una riforma sgangherata della Costituzione che è stata bocciata senza appello dal voto del 4 dicembre: una darà le carte da palazzo Chigi e l'altra interpreterà il ruolo di Ministro per i rapporti con il Parlamento. C'è nel suo Governo lo stesso Ministro che sosteneva che il lavoro dei giovani è oggi meno precario e più stabile e i giovani hanno risposto con il loro voto il 4 dicembre. Non c'è, è vero, la ministra Giannini perché anche Renzi aveva capito che la cosiddetta buona scuola non era affatto buona prima di imporre la fiducia, lo aveva convinto il senatore Tocci, eppure ha comunque imposto la fiducia perché alcuni *pasdaran* gliela hanno chiesta.

Il voto del 4 dicembre è un po' come il voto sul divorzio, chiude un mondo e lo cancella: il mondo in cui si pensava ci si dovesse affidare ad un solo uomo al comando, il mondo in cui si cercavano leggi maggioritarie, in cui si sceglieva tra democratici e repubblicani, mediati e moderati al centro dal ceto medio. Quel mondo è scomparso, perché dal 2008 in poi la crisi ha spazzato via

il *referendum* indica la strada su cui procedere, per realizzare questo confronto in Parlamento, che anche lei dice di volere, quella di cancellare la legge Italicum, che è stata imposta con tre voti di fiducia dal Governo Renzi, e riscriverne una che abbia due caratteristiche fondamentali: la prima è il no a premi truffa, che trasformino una minoranza nel Paese in maggioranza parlamentare; la seconda è quella di ridare agli elettori il diritto di eleggere gli eletti. Ci sono molte possibilità per attuare queste due indicazioni di fondo, che vengono dal corpo elettorale: discutiamone. Trovo che in questo Parlamento si stia cominciando a discutere, trovo vi sia la possibilità di parlare in modo franco e produttivo,

Aspettiamo che ci faccia delle proposte e, anche quando sono dolorose, la invitiamo a dire la verità, a non dissimulare, a non usare i toni della propaganda, ma il confronto. Opposizione non significa guerra, ma dare un contributo per il bene del Paese. Signor Presidente, signori Ministri, signor presidente Gentiloni ho letto e apprezzato le sue dichiarazioni programmatiche, che evidenziano sostanzialmente la sua buona volontà dimostrare un impegno ad affrontare questioni che hanno pregnanza sia sul piano formale, che sostanziale. Apprezziamo soprattutto la sobrietà dello stile, che ci fa sperare e che riteniamo utile perché si riprenda nel Paese un dialogo costruttivo che porti verso una pacificazione del quadro politico, tanto anelata quanto difficile, perché ostacolata da forze politiche, che alimentano il proprio consenso sulla debolezza delle istituzioni dopo la vittoria del no al *referendum* e sulla crisi sociale ed economica, che purtroppo attanaglia la nostra Nazione. Queste forze politiche, proprio nel momento in cui, prima di ogni altra cosa, avremmo la necessità di metterci intorno ad un tavolo per scrivere regole condivise, spostano i problemi sulla piazza, per infuocare lo scontro sociale, facendo leva su un oggettivo malessere, che la crisi economica, che si protrae da anni, ha purtroppo determinato. Noi invece, presidente Gentiloni Silveri, abbiamo pensato che la maniera migliore per rispondere alle difficoltà in cui versa in questo momento l'Italia sia un forte richiamo alle nostre coscienze, per un'ulteriore assunzione di responsabilità, che possa contribuire a far uscire il nostro Paese dalla palude istituzionale in cui si trova. In quest'ottica abbiamo apprezzato le scelte del Capo dello Stato e abbiamo dato la disponibilità ad appoggiare un Esecutivo, che non è, come qualcuno ha detto, un Esecutivo di sopravvivenza ma un Governo a tutti gli effetti che ha il difficile compito di traghettare l'Italia verso una nuova fase di democrazia e di partecipazione attraverso la costruzione di regole che garantiscano governabilità e credibilità internazionale al nostro Paese. Noi ci riconosciamo nei metodi e nelle intenzioni del nostro Presidente della Repubblica, nel suo senso delle istituzioni, nella necessità di avere una riforma elettorale che sia omogenea e armonica tra le due Camere per garantire governabilità. Questo - sia chiaro - non è un pretesto per fare andare avanti una legislatura che a qualcuno può sembrare logora o consunta, ma è un ragionamento che deriva dalla consapevolezza che consegnare agli italiani un Parlamento con due Camere elette con sistemi elettorali diversi - maggioritario alla Camera e proporzionale al Senato - è, a mio avviso, un attentato alla governabilità e alla democrazia rappresentativa. Non abbiamo scadenze o date da traguardare. Non abbiamo obiettivi temporali, ma abbiamo un programma che ci siamo impegnati ad appoggiare già da tre anni e che necessita di essere completato, nel segno della continuità con il precedente precedente Governo, che ha avuto un'interruzione traumatica di un percorso positivo, virtuoso, segnato da una lenta ma sicura ripresa, da un tentativo faticoso di uscire da una crisi che si protrae da tempo. La continuità, che per qualcuno è un limite, dal mio punto di vista è un valore aggiunto; è il risultato di tre anni di impegno da parte di un Governo che ha rimesso in moto il Paese, e noi siamo orgogliosi di avere appoggiato questo percorso. Guai, però, a pensare che la legge elettorale sia l'unica emergenza di questo Paese. Incombono alcune scadenze, nodi non risolti, *dossier* aperti che hanno urgenza di essere definiti; non soltanto la crisi del Monte dei Paschi e del sistema bancario con più di due milioni di correntisti in ansia per ciò che sta accadendo, di una rete economica che viene tenuta insieme dal sistema bancario. Il suo Governo, signor Presidente, dovrà occuparsi di altro: di adottare misure per far fronte all'emergenza terremoto; di pensare all'attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale; della definitiva applicazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza che, grazie all'impegno del ministro Lorenzin, finalmente sono stati riesumati dopo anni e anni che sono stati tenuti nel cassetto. Dovrà attuare misure di contrasto alla povertà, *jobs act* autonomi, la riforma dei *voucher* per evitare forme di abuso sul mercato lavoro. Signor Presidente, se voi ritenete che anche la riforma del processo penale sia un'urgenza, che ben venga, però è bene che si sappia che da parte di questo Gruppo politico non c'è alcuna volontà o voglia che questa riforma, che viene fuori dopo sei o sette mesi di discussione nella Commissione giustizia

Infine, ma sicuramente non ultima, signor presidente Gentiloni Silveri, c'è la salvaguardia occupazionale dei lavoratori precari siciliani. Glielo dico da siciliano, ma lo dico perché riguarda 20.000 lavoratori, 20.000 famiglie, che dal 1° gennaio 2017 rischiano per la prima volta, dopo più di vent'anni, di restare senza stipendio. Rischiamo una vera e propria esplosione sociale; un'emergenza in una Regione che, secondo gli ultimi dati ISTAT, è la più povera d'Italia. A questo proposito dobbiamo esprimere il nostro apprezzamento per l'istituzione del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, perché proprio da quella parte dell'Italia deve arrivare una spinta forte per accelerare la ripresa economica e ridurre il differenziale, il *gap*, tra le due parti del Paese che lo vedono sempre più spaccato in due. due. Signor Presidente, noi siamo felici di appoggiare un Governo da cui pretendiamo una coda di legislatura improntata al senso di responsabilità, al pragmatismo, a fatti concreti, allo sforzo vero di restituire all'Italia un'effigie di unità nazionale. Credo che lei e la squadra che ha formato sarete in grado di operare al meglio, nonostante il poco tempo a disposizione. Buon lavoro a tutti voi. signor Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, ricordiamo tutti la scena dell'allora presidente del consiglio Renzi che si presentò in quest'Aula del Senato, con tono spavaldo e la mano in tasca, per dire che chiedeva la fiducia a questa

Siamo qui per la fiducia, che il Gruppo di Forza Italia non le darà, ma ovviamente non possiamo non parlare delle macerie in cui lei si trova, perché Renzi le ha lasciato una serie di polpette avvelenate. È quel Renzi che disse che si sarebbe ritirato a vita privata: non sappiamo se lo farà, per ora ha preso atto che il 60 per cento dell'Italia gli ha votato contro, ma ricordiamo tutte le frasi roboanti per cui lui sarebbe tornato a fare il cittadino comune se avesse perso al *referendum* che lui si è intestato, con tutte le conseguenze che abbiamo visto.

San Matteo del 2014: o hanno abolito San Matteo o non hanno rimborsato questi debiti. Ho l'impressione che il Santo rimanga nelle liturgie, ma anche i debiti non pagati. Non parliamo poi del Sud, che adesso è affidato alle cure taumaturgiche di un Ministro e chissà se ricomparirà nell'agenda della politica. presidente Gentiloni Silveri, di cui parlerò tra qualche momento nelle mie conclusioni. Il presidente Renzi ha lasciato in maniera irresponsabile una polpetta avvelenata: ha varato una legge elettorale per la Camera e volutamente non per il Senato, con un atteggiamento irresponsabile che priva il Presidente della Repubblica del legittimo potere di mandare gli italiani

oggi che è Presidente del Consiglio. Si ricordi del suicidio delle sanzioni alla Russia che danneggiano la nostra economia. È ora di finirla: Obama non c'è più. Non prendiamo più ordini sbagliati dagli americani, oltre tutto Putin nei confronti del terrorismo fondamentalista ha dimostrato più coraggio e idee chiare

nel Paese. Abbandonate poi la presunzione. Avete piegato organizzazioni di categoria - i cappellini gialli della Coldiretti - e divulgato dati fasulli della Confindustria per spaventare il Paese e incoraggiare il sì. C'è stata anche un'azione di condizionamento delle associazioni di categoria che dovranno risponderne ai loro associati, che non hanno votato

dimostra che la politica non si improvvisa. Lo dica a qualche suo Ministro che non conosce l'abc della politica e ha fatto più anni di Governo che di militanza politica. L'improvvisazione in politica è un altro errore del Governo Renzi; almeno con lei l'improvvisazione certamente non c'è. Anche il senatore Zanda e tanti

Renzi. Questi sarebbe ancora al suo posto se non avesse avuto la presunzione di mandare in Europa la Mogherini invece di D'Alema e se avesse mantenuto il rapporto leale con Berlusconi che, nonostante le amarezze e le ingiustizie patite e anche l'applicazione illegittima e retroattiva della legge Severino, mantenne un patto sulle riforme fino a quando l'arroganza di Renzi

(noi abbiamo grande rispetto per il Presidente della Repubblica) contestammo il metodo dell'imposizione, non la qualità delle persone. Lei questi errori non credo lì farà per il tempo che dovrà governare. Non vedo i colleghi del Gruppo ALA-Scelta Civica Su di loro grava il fattore «t», presidente Gentiloni Silveri. Loro sono stati «leali» con Renzi e la sinistra, però voi li avete considerati «letali» per il vostro Governo: c'è una «t» in aggiunta che da leali li fa diventare letali.

poi ci sono gli altri giorni. Il Senato non è stato abolito, ha i pieni poteri, può dare la fiducia, approva tutte le leggi. Non si illuda. Quindi, sulla legge elettorale si confronti con la democrazia e con il Parlamento e, per il resto, corregga gli errori. Per l'immigrazione lei sta per andare in Europa, ma il problema non è

Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Presidente del Consiglio e Governo, permettete una prima breve osservazione di metodo: capisco tutte le scadenze e le urgenze, compresa quella obbligata di domani in Europa. Però, in generale per il futuro, e se possibile, consiglierei meno fretta, meno corsa e più tempo di ponderazione e pause di riflessione. Mi soffermerò soltanto su un punto, signor Presidente quel passaggio delle sue comunicazioni alle Camere, dove riconosce - gliene do atto - che su due grandi problemi non ci sono state, nell'immediato passato, risposte sufficienti: l'area sociale della parte più disagiata della popolazione e l'area territoriale del Mezzogiorno. Considero una scelta opportuna aver concentrato in un Ministero la cura di questi problemi ritengo rassicurante la competenza e la professionalità del ministro De Vincenti, ma qui c'è un tema enorme che chiede di essere affrontato, e, direi, aggredito in grande. Non è tema solo per noi, ma lo è per l'Europa e per l'intero Occidente. Irrompe e ci interroga una nuova questione sociale, inedita per la sua composizione materiale e per i modi della sua espressione formale; viene da lontano, e la colpa della politica, o delle politiche, è di non averla vista arrivare: grave colpa. La mutazione del capitalismo, dalla struttura storica a centralità dell'industria manifatturiera verso un "finanz-capitalismo" e un "ordoliberismo", per un po' è stato il nuovo che avanzava e per due decenni ha potuto vivere della spinta propulsiva, fatta di sviluppo economico e innovazione tecnologica; poi, fatalmente, ha visto incepparsi il meccanismo di crescita ed è precipitato in una crisi lunga, profonda, diffusa, globalizzata dalla stessa globalizzazione in atto. La crisi ha messo a nudo le sue contraddizioni e le ha scaricate sul basso del sociale, frantumando le appartenenze tradizionali e disordinando quella coesione orizzontale che la società industriale divisa in classi aveva a suo modo assicurato. L'inedito del blocco sociale che si è ricomposto vede l'emarginazione del lavoro dipendente e la svalorizzazione del lavoro autonomo, di varia generazione. È, sì, questione di reddito, di stabilità del lavoro, di assicurazione del futuro, ma è questione anche (e di questo si tiene poco conto, perché manca alla politica la psicologia di massa) di *status*. L'operaio di Detroit o di Torino, con la sua alta cultura industriale, di fabbrica, non sopporta, non accetta, di diventare un emarginato sociale. Il ceto medio, che abitava il luogo di un ascensore sociale che saliva, non sopporta e non accetta di vederlo scendere, trascinandolo a una condizione di semiproletarizzazione. Di qui, la reazione aspra, che si esprime nella rabbia contro tutto e contro tutti. È questa la base materiale, strutturale, dello strappo che si è realizzato tra cittadini e istituzioni, tra massa ed *élite*, tra le persone in carne ed ossa e i cosiddetti politici virtuali, tra popoli e Governi. Se non si sana questo strappo, se non si ricostruisce chirurgicamente questo legamento, non è possibile né un Governo efficiente, né un'opposizione responsabile. Vorrei dirlo a questi banchi vuoti, a memoria futura, e a quelle forze di movimento che credono di utilizzare questa criticità in funzione di un immediato consenso: non insistete ad attizzare questo fuoco, perché ne rimarrete anche voi bruciati. Andando al governo in queste condizioni, dopo qualche mese sarete voi l'*élite* contro cui si scaglia la massa, sarete voi l'*establishment* combattuto dai cittadini. Questo, quindi, è un problema da risolvere in precedenza, è la *condicio* per l'agire politico di chiunque. Questa storia della pancia e della testa andrebbe allora forse messa in ordine. chi parla alla pancia e chi parla alla testa. Io direi così: dare attenzione con la testa alla pancia del Paese; il che vuol dire una cosa semplice, oggi però difficile da praticare: interpretare politicamente il disagio sociale e curare con la politica, non con l'antipolitica (anzi, contro l'antipolitica), la sofferenza di chi sta male. Dall'alto delle istituzioni, Parlamento e Governo devono piegarsi umilmente verso terra per vedere quello che c'è nel basso del sociale, il malessere, il rifiuto, il rancore, a volte malamente spesi, ad esempio contro gli immigrati, o con altri diversamente poveri, per andare a colpire i motivi veri e reali, che spesso si riducono a uno solo: la quotidianità insopportabile di una vita senza dignità. Colleghi, siamo qui per questo; noi a rappresentare, voi a governare. Presidente, forse il suo Governo non potrà fare molto, se non altro per i tempi assegnati, ma alcuni segnali e alcuni paletti possono essere dati e messi. Mostrare un'intensa sensibilità su questo versante sarebbe già qualcosa di nuovo. Concludo, presidente Grasso. Non so o non ho capito che cosa sia questa cosiddetta *post-*verità. So che una volta si affermava che «dire la verità è un atto rivoluzionario»; non sì può dire più, purtroppo (e sì che mi piacerebbe), ma è meglio dire la verità che spargere illusioni. dire, ad esempio: questi sono i problemi, li conosciamo, li pratichiamo, i margini sono stretti, le cose fatte in passato pesano, le compatibilità nazionali e sovranazionali premono, nel risolvere i problemi la volontà deve fare i conti con il tempo necessario per fare bene. È vero - ed è stato già osservato - che si è creato un contrasto, attraverso il quale è passato, a mio parere (forse sbaglierò), parte consistente del no che ci ha punito in questi giorni, tra la narrazione sulla condizione del Paese Italia e la percezione della stessa condizione da parte di milioni di persone; narrazione, da un lato, e una percezione, dall'altra, in conflitto. Ecco, su questo punto non invoco una discontinuità, ma consiglio una correzione di accento. Responsabilizzare i cittadini è il modo migliore per convincerli, chiamarli a collaborare a una missione comune: si guadagna in serietà, in credibilità, in affidabilità; in serietà, in credibilità, in affidabilità; le doti che l'uomo di governo deve faticosamente e con pazienza mostrare di possedere, giorno dopo giorno. Buon lavoro

La seduta è ripresa.

colleghi che è in corso la trasmissione diretta televisiva con la RAI. Ha facoltà di intervenire in replica il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gentiloni Silveri. Signor Presidente, onorevoli senatori, signore Ministre e signori Ministri, nel rivolgermi al Senato per chiedere la fiducia al nuovo Governo ci sia un punto di partenza obbligato. Voi sapete che io ho condiviso

certamente basata sull'articolo 94 della Costituzione, ma è anche un po' particolare: chiedo la vostra fiducia ed esprimo la mia fiducia nei confronti del Senato

Io credo che le cose siano molto chiare e lo siano anche per i cittadini italiani. Si è dimesso il Presidente del Consiglio, si è aperta una crisi di Governo. E penso che la scelta del presidente Renzi di dimettersi, in coerenza con quanto aveva ripetutamente annunciato nel corso della campagna referendaria, sia stata una scelta di coerenza che merita il rispetto di tutti coloro che hanno a cuore la dignità e la serietà della politica. Si possono fare tutte le polemiche che vogliamo, ma vi è il dato di fatto di un Presidente del Consiglio che, pur disponendo ancora di una maggioranza e quindi non essendo obbligato in termini formali e costituzionali, sceglie di dimettersi. Non siamo innamorati della continuità. Abbiamo, anzi, rivolto una proposta all'insieme delle forze parlamentari per individuare, se possibile, una convergenza più larga, addirittura una convergenza generale di fronte alla situazione. è stata da parte della stragrande maggioranza delle forze politiche a cui questo invito era stato rivolto una indisponibilità. Quindi non un amore per la continuità, ma la presa d'atto di questa situazione ha spinto le forze che hanno sostenuto fin qui la maggioranza a dare vita al nuovo Governo, per responsabilità, come ho cercato di sottolineare ripetutamente in questi giorni. Sarebbe stato forse più utile dal punto di vista politico e partitico - se volete - sottrarsi a questa responsabilità, ma sarebbe stato molto più pericoloso per il Paese. Pertanto, il segno di questo Governo è di farsi carico di questa situazione. Molti hanno parlato di verità anche se forse come diceva il senatore professor Tronti - la verità rivoluzionaria non è più di moda, ma questa è la verità: che il Governo si è costituito con queste caratteristiche per assumersi una responsabilità che riteniamo fondamentale in questo momento. Lo abbiamo fatto in modo molto rapido: nove giorni fa il *referendum*, una settimana fa le dimissioni del presidente Renzi, due giorni fa l'incarico al sottoscritto di formare un nuovo Governo; non per impazienza, ma perché credo sia a tutti evidente l'importanza di dare all'Italia istituzioni stabili e certezza, in un contesto come quello attuale. infatti, che abbiamo impegni immediati sui quali il Governo è al lavoro e sarà al lavoro con ancor più forza nella pienezza delle sue funzioni. Penso al sostegno al sistema bancario, di cui ho parlato anche nelle mie comunicazioni iniziali. Penso all'emergenza terremoto e ricostruzione: sarà la prima riunione che farò oggi pomeriggio con il commissario Errani e con il direttore della Protezione civile. Penso all'impegno europeo: domani mattina vi è un Consiglio europeo in cui è importante che l'Italia sia rappresentata a pieno titolo, perché si discuteranno alcuni temi molto rilevanti, come le regole sui flussi migratori, in particolare sui rifugiati, in merito alle quali voi conoscete la posizione italiana, quindi non la ripeto.

Grazie, dei maggiori non successi - purtroppo - della diplomazia internazionale e, per la parte che compete all'Italia, del sottoscritto negli ultimi mesi. È stata una partita nella quale abbiamo cercato di sperimentare anche nuovi rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia; per un certo periodo sembrava che questi nuovi rapporti tra Russia e Stati Uniti per arrivare a una tregua purtroppo questo non si è sviluppato e continuiamo ad assistere a un dramma che offende le nostre coscienze e che l'Assemblea del Senato credo debba ricordare come una tragedia inaccettabile per la nostra civiltà. Rinvio alle comunicazioni che ho fatto all'inizio per una serie di impegni serie di impegni programmatici che attendono il Governo. Questo non è un Governo di inizio legislatura, ma è un Governo che innanzitutto deve completare l'eccezionale opera di riforma, innovazione e modernizzazione che è stata fatta in questi ultimi anni. non c'è dubbio, io credo. Si possono avere opinioni diverse e si possono naturalmente, dal punto di vista dell'opposizione, più che legittimamente criticare molte di queste riforme e di questi cambiamenti:

e sarebbe assurdo che un Governo, che peraltro molti tra i critici accusano di eccesso di continuità, immaginasse che completare il percorso di riforme avviato non è il suo compito principale. Quindi giustizia, diritti, completamento delle norme sulle pensioni, innovazione (mi ha colpito il riferimento che vi ha fatto la senatrice Cattaneo nel suo intervento) e un accento particolare, che io ho voluto dare sin dalle comunicazioni iniziali, al tema del lavoro e del Sud. è uno dei luoghi nei quali contemporaneamente si manifesta la maggiore potenzialità del nostro Paese, perché, se il nostro Paese può avere nei prossimi anni un tasso di crescita molto più alto di quello attuale, ciò sarà possibile se riusciremo a fare molto di più per il Mezzogiorno. Non abbiamo in testa chissà quali operazioni all'antica, quando parliamo di un Ministero che ha tra le sue competenze il Mezzogiorno; tutt'altro, abbiamo in testa la straordinaria opportunità che, se impostiamo bene questa partita, può venire da una rinascita e da una ripresa del Mezzogiorno. Lavoro e Mezzogiorno (Mezzogiorno continentale e insulare) sono tenuti insieme dal tema che il senatore Tronti ha affrontato; chiamiamolo il tema del disagio che oggi si accompagna con gli sviluppi e con i progressi della modernità. Voi sapete bene che siamo contemporaneamente in uno dei momenti più felici dell'umanità, perché questo è uno dei momenti nei quali la vita media si è più allungata, la capacità di contrastare le malattie si è rafforzata, ciascuno di noi ha nelle proprie tasche una quantità di conoscenze incredibile, che solo per la mia generazione avrebbero reso necessarie biblioteche intere, cui noi possiamo accedere invece con grandissima semplicità (poi c'è anche la velocità dei trasporti). Eppure, di fronte a questa straordinaria evoluzione della modernità, c'è, in modo particolare nelle società occidentali, libere e avanzate, un problema crescente di disagio in alcuni strati e in alcune fasce sociali. Sono in particolare le fasce più deboli e più povere del ceto medio quelle che stanno sentendo in modo pesantissimo le conseguenze di questi fatti positivi, del fatto che il mondo è più aperto e del fatto che l'evoluzione tecnologica è più forte. Se qualcuno pensava a questo mondo più aperto e a questa evoluzione tecnologica più forte come ad una sorta di nuovo Ballo Excelsior - e lo abbiamo pensato in molti negli ultimi dieci-quindici anni - si sbagliava di grosso. Certamente c'è uno straordinario progresso, ma ci sono le difficoltà, il disagio, i perdenti in questo processo e a chi a questo processo tiene, cioè a chi è innamorato dell'idea della società aperta

da questi grandi progressi invece è colpito, subisce conseguenze pesanti, addirittura vive peggioramenti della propria situazione. Ci sono dei dati resi noti stamattina dal centro studi della Confindustria che sono da questo punto di vista molto interessanti. Da una parte, infatti, fanno vedere una cosa che è sotto gli occhi di tutti e che, in buona misura, è anche il risultato dell'azione svolta svolta in questi ultimi anni, cioè, che i tassi di crescita vengono previsti con un rialzo maggiore delle previsioni e che c'è più crescita di quanto si prevedeva I tassi di disoccupazione vengono, sia pur molto lievemente, proiettati più bassi di quanto si prevedeva. Si tratta quindi di dati macroeconomici incoraggianti, che fanno vedere che l'Italia si è rimessa in moto, che in Italia e in Europa c'è, lentamente e gradualmente, un segno di ripresa. Al tempo stesso avete però visto nei dati resi noti dal centro studi della Confindustria quelli sulla povertà, sulla povertà, che sono anch'essi in crescita. Ci dobbiamo rendere conto di questa contraddittorietà del contesto in cui siamo e in cui sviluppo, progresso, modernizzazione, convivono con sacche di disagio

Questo è il senso della sottolineatura particolare; non abbiamo vent'anni davanti per cambiare il volto al Mezzogiorno d'Italia, ma è il senso della sottolineatura particolare della parola Sud e della parola «lavoro, lavoro, lavoro», che ho cercato di fare in questi giorni. Cercheremo di lavorarci con serietà, approfondendo anche la questione dei tempi e dei modi possibili di procedere verso l'universalizzazione delle tutele,

percorribile con serietà e consapevolezza perché non lo risolviamo purtroppo con facili *slogan*. Ho parlato nelle mie comunicazioni introduttive della durata del Governo, che è stabilita dalla Costituzione. Ho parlato della legge elettorale, rispetto alla quale rivendichiamo un compito di

comunque, a prescindere da quanto durerà o non durerà la legislatura, l'urgenza di dare al nostro sistema regole che consentano di votare alla Camera e al Senato in modo armonizzato ed effettivo. Questa è un'esigenza del del sistema e delle istituzioni. Non è una valvola da aprire o chiudere a seconda dell'urgenza o minore urgenza dell'appuntamento elettorale. Per questo dico che il Governo non sarà attore protagonista, sarà facilitatore e solleciterà

influenzerà, in parte, perfino la costituzione materiale del nostro Paese, come si suol dire, perché credo che sia giusto il riferimento, che leggiamo sui giornali e che qui è stato ripreso da alcuni colleghi da Quagliariello e da Mineo, anche se su fronti opposti, sul fatto che non vi è dubbio che in gioco vi sia anche l'evoluzione del nostro sistema rispetto a come è stato negli qui mi fermo perché, nel mio ruolo attuale, non posso andare oltre ma non vi è dubbio che quando discuterete - e il Governo darà il suo contributo le nuove regole elettorali, saremo tutti consapevoli che si tratterà di una discussione che incederà sul modo di concepire il funzionamento della nostra democrazia. Questo credo sia un aspetto di cui certamente tenere conto. Io difenderò, com'è ovvio, le prerogative del Parlamento e lo farò nei confronti di tutti. C'è stata una discussione a mio parere molto sbagliata negli ultimi mesi da parte di chi ha presentato le riforme che erano state approvate, peraltro a maggioranza, nel Parlamento come chissà quale tentativo autoritario. Credo che questo sia stato un errore. Invito, comunque, chi, in questi mesi, si è battuto alzando la bandiera del Parlamento contro ipotetici e - a mio avviso - inesistenti, tentativi autoritari, a rispettare il Parlamento e le sue regole, a partecipare alle sue riunioni e a farlo in modo civile e dignitoso come prevede la Costituzione.

Chiedo a tutti i Ministri del Governo che ho l'onore di presiedere di lavorare con responsabilità e con dignità. Aggiungo solo un'altra parola che rubo ad un grande italiano, il presidente Ciampi, un grande statista italiano, che quando presentò, in tutt'altre condizioni, il suo Governo, usò un altro termine molto importante, il termine «umiltà», e disse

in matematica ci sono tre specie di discontinuità: di salto, essenziale, eliminabile. Quella essenziale è la discontinuità per eccellenza, dove non è possibile ricondurre la funzione ad un unica visione continuativa e uniforme. Avremmo voluto una discontinuità essenziale di questo Governo, vista l'essenzialità del risultato referendario: è un volere non mio, ma di milioni di italiani. Qui ci troviamo di fronte ad una discontinuità non essenziale, ma ad una discontinuità eliminabile, dove il puntino che oggi manca alla funzione governativa è solo il piccolo, piccolo Matteo. Noi, cordialmente, a Gentiloni Silveri dovremmo dare la fiducia? Diciamo no a questo punto di discontinuità, no a tutti i "rim-Boschi-menti", no a tutti i "comp-Lotti". Noi del Movimento X valuteremo la possibilità di una fiducia, quando vedremo eliminati, per coerenza, coloro che hanno promesso di andarsene, quando vedremo discontinuità essenziale e, soprattutto, quando vedremo approvata la legge sul *care giver*, ovvero il familiare assistente, invece di vedere al Governo assistenti di familiari. rappresentanti del Governo, tenendo fede a quanto riferito nel colloquio con il presidente della Repubblica Mattarella, in merito ad un Governo che consenta in tempi congrui il voto agli italiani, previa legge elettorale omogenea, che assicuri rappresentatività e governabilità, e che nelle more lavori per dare risposte alle emergenze del Paese, prendiamo atto della nascita e della composizione del Governo che lei, signor presidente Gentiloni Silveri, oggi viene a proporre al Senato. Per responsabilità istituzionale le assicuriamo la fiducia da parte dell'Italia dei valori. Seguiremo con attenzione l'attività e i provvedimenti che porterà in questo ramo del Parlamento, che per volontà popolare è rimasto centrale nella vita istituzionale e politica del Paese. Ci renderemo promotori e ci adopereremo affinché vengano posti al centro dell'azione del nuovo Governo temi a noi cari, come la riforma dell'istituto della legittima difesa, da noi proposta attraverso una legge di iniziativa popolare, su cui sono state raccolte più di due milioni di firme,

motorie, e perseverare sulle politiche di inclusione sociale, per diminuire le diseguaglianze, portando milioni di persone fuori dalla situazione di povertà. Concludo con ultimo punto, che è tale solo nel decalogo, ma non per valenza: signor Presidente, la esortiamo a rispettare il suo lavoro attraverso le politiche sul e per il lavoro - per i nostri giovani e non - e per il rilancio del Sud del Paese. Contribuiremo, per senso di responsabilità, con la nostra partecipazione alla nascita di questo Governo, riservandoci di assicurare il nostro sostegno in base alle risposte che il nuovo Esecutivo darà ai temi a noi cari. non possiamo che augurarle e augurarci un buon lavoro, per l'Italia e per gli italiani, affidandole questa apertura di credito da parte dell'Italia dei valori. signor Presidente del Consiglio, colleghi, questo Governo nasce in seguito alle dimissioni del presidente Renzi, che non erano affatto dovute, come ha detto il presidente Gentiloni, che sono il risultato di un atto di coerenza raro - anzi unico, se vogliamo - nella vita politica italiana e che dunque va apprezzato o almeno rispettato. Renzi aveva preso sul serio il mandato ricevuto dall'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano di trasformare questa legislatura, che era nata zoppa, in una legislatura costituente e così ha portato avanti la riforma costituzionale, che è stata poi varata dal Parlamento e che poi, come sappiamo, è stata bocciata dal popolo italiano - ahimè - con un voto politico e non di merito. Tale risultato ovviamente va comunque rispettato, anche se resto convinta che sia stato un errore bocciare questa riforma, che era necessaria per modernizzare le istituzioni. Renzi e gli alleati di Governo, primo tra tutti il ministro Alfano, hanno avuto il merito di battersi per il cambiamento, sfidando l'immobilismo, il conservatorismo e l'irresponsabilità di molte forze politiche. La strada del cambiamento oggi non ha alternative e non può averne, se non vogliamo rassegnarci alla decadenza del Paese. La revisione delle legge elettorale sarà un importante banco di prova, se non del Governo, comunque della maggioranza e di quelle forze politiche che si sono rese disponibili a discuterne. Presidente Gentiloni sono certa che lei proseguirà sulla strada delle riforme e che farà un buon lavoro, aiutando il Paese a uscire da questa crisi sociale e politica. Concludo, signor Presidente, dicendo che, con questo spirito mi accingo a votare con convinzione la fiducia al suo Governo

Non ho alcun motivo per ringraziarlo sul piano personale, ma sul piano politico come cittadino lo ringrazio per due motivi. Ha mostrato coraggio nel battersi per il cambiamento ed è stato all'inizio un buon *coach*: ha saputo infondere in noi cittadini un senso di orgoglio, di appartenenza, di speranza. Grande tecnico, in particolare della comunicazione e della motivazione, ha finito, purtroppo, per la sua inadeguatezza politica, con il recare danno al Paese. Si è risolto, purtroppo, in un danno aver scelto come priorità assoluta la riforma della Costituzione, finalità importante e nobile, ma condotta in modo non soddisfacente. Si è risolto in un danno, nella calibratura specifica della riforma, avere sottovalutato l'importanza che avrebbe avuto allargare ulteriormente il consenso nel Parlamento

che però si è realizzata - della Costituzione della Repubblica italiana, riguardante l'articolo 81 (e non, come si dice, il *fiscal compact*), l'allora ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda fece, con umiltà, un attentissimo lavoro che portò ad avere il 73 per cento di voti favorevoli in questa Camera

Chi le parla, signor Presidente del Consiglio, è stato iscritto in un nuovo raggruppamento, chiamato «della accozzaglia». mi sono speso doverosamente nell'interesse del Paese, in questi ultimi mesi, per spiegare, soprattutto all'estero, che, a mio giudizio, erano completamente fuori luogo le previsioni, alimentate anche dall'Italia e da quegli ambienti finanziari internazionali dei quali si è a lungo detto che io ne sarei controllato, e che stavano grossolanamente sbagliando. Anche in caso di vittoria del no non ci sarebbe stato né un cataclisma finanziario

per la fiducia che ho in lei e in diversi suoi Ministri. È una fiducia condizionata a tre linee di condotta che auspico di vedere realizzate. Per quanto riguarda l'Europa, materia che lei conosce così bene, che alla sostanziale povertà di risultati, ma altezza di toni, si faccia seguito con una politica molto più incisiva e meno inutilmente rumorosa. Per quanto riguarda l'economia, ho totale fiducia nel ministro Padoan e voglio pensare che, in questo periodo così laboriosamente orientato dal Capo del Governo alla finalità *referendum*, qualche volta non abbia fatto tutto ciò che avrebbe ritenuto ottimale lui stesso fare. Abbiamo perso tempo per la crescita, per il consolidamento fiscale, per le banche, e sono sicuro che il vostro Governo darà grande priorità a questo. condizione che osserverò in futuro per orientare il mio voto sui singoli provvedimenti e il mio apprezzamento del Governo riguarda semplicemente la serietà. Mi auguro

che si sostituisce al sereno e anche aspro confronto sulle opinioni e mi auguro di non vedere più toni sprezzanti che nuocciono al Paese e a chi li pone in atto. Tra le priorità ho ascoltato con molto interesse l'intervento del senatore Tronti. Se vogliamo stare sulla verità e non sulla post-verità, credo che il tema delle diseguaglianze e una politica per una

un Esecutivo che in 1.000 giorni pone la fiducia 63 volte non rispetta la Costituzione, marginalizza l'attività del Parlamento e cambia le regole del gioco democratico. Parta da questa considerazione, presidente Gentiloni Silveri: la seguiremo con attenzione e parteciperemo con lealtà e con rigore al percorso che di qui alle imminenti - vogliamo sperare - elezioni politiche accompagnerà l'azione del suo Governo, innanzitutto nel ripristino delle condizioni della democrazia parlamentare. Si detto, anche da parte di colleghi intervenuti in questo dibattito, che il Paese è lacerato. È vero e forse i livelli della lacerazione sociale sono diventati addirittura più imponenti e impellenti rispetto alle difficoltà economiche, alle disuguaglianze, alle contrapposizioni che si sono determinate per un'assoluta e totale inefficacia dell'azione politica. Io non so, signor presidente Gentiloni, quanto il massiccio voto negativo alla riforma costituzionale tragga origine dalle motivazioni di un dissenso sul contenuto di quella riforma e quanto invece sia il frutto di un metodo di lavoro che gli italiani non hanno apprezzato. Infatti, quando nella politica la disciplina di partito prevale sul dibattito, quando la prepotenza del Governo irrompe nell'autonomia del Parlamento, quando l'arroganza del potere prevale sulla capacità di ascolto e di mediazione alta tra le differenti posizioni e sensibilità, a patirne non è un partito politico, ma la democrazia; il Paese, con il suo voto e con la sollevazione popolare, ha voluto dare una indicazione netta, precisa ed inequivoca alle forze politiche, al Governo e al Parlamento. Questo è il risultato della consultazione referendaria, signor presidente Gentiloni Silveri. Noi Conservatori e Riformisti non amiamo né i toni alti, né le polemiche, né le urla; noi cerchiamo di attingere al nostro modesto patrimonio di propositività per dare indicazioni, non omologandoci alle strumentalizzazioni politiche, ma volendo partecipare con onestà intellettuale, con coerenza e lealtà alla formazione delle leggi che servono al Paese. In tal senso non tradiremo la nostra azione e il nostro impegno, come dimostrato in questi anni con la schiena dritta e con grande rispetto e determinazione.

a casa - acclarasse ed evidenziasse ancora di più le conseguenze e le determinazioni successive. È vero che ci sono state le dimissioni, però, presidente Gentiloni, mi permetta di dirle che il Paese non ha gradito - e certamente non lo abbiamo gradito noi - vedere il presidente Mattarella, con la sacralità di un ruolo interpretato in modo impareggiabile,

della senatrice Rizzotti)*. Non si era mai visto che un Presidente dimissionario avviasse contestualmente alle consultazioni del Capo dello Stato delle consultazioni a Palazzo Chigi. Mi permetta di dirle

con un Governo che sa già di vecchio, con un Governo che oggi assume una responsabilità che, sinora, non sembra marcare una discontinuità rispetto al passato.

Propaganda e mancette, pannicelli caldi e un'arma di distrazione di massa, qual è stata la lunga campagna referendaria con l'occupazione dei servizi pubblici radiotelevisivi, governo quali le politiche sociali, lavoro, pensioni, assistenza, politica economica e fisco, crisi del sistema bancario, Monte dei Paschi di Siena, sicurezza dei territori, politica estera tra Europa e crisi siriana.

di cui ci ha parlato e il rispetto che vorrà destinare alle Aule del Parlamento, riportando equilibrio e pacificazione tra i poteri costituzionali, rappresenteranno condizioni adeguate e sufficienti per consegnare destini diversi all'impegno che con Raffaele Fitto, come Conservatori e Riformisti, abbiamo profuso in questi anni, quando abbiamo registrato supponenza e indifferenza finanche davanti a proposte emendative di buonsenso finanziate e strutturate, come il tetto fiscale in Costituzione e la perequazione infrastrutturale Nord-Sud.

un'azione di governo capace di recuperare nell'agenda dell'Esecutivo un efficace contrasto all'emarginazione di un'intera area del Paese. Credo che la demagogia di

della sicurezza e della legalità dei territori, dei servizi pubblici. Ma il Mezzogiorno - come ben sa il professor Claudio De Vincenti - è anche ILVA, è anche Taranto, con quelle genti dimenticate che ancora continuano a morire, dove un emendamento di cinquanta milioni di euro per finanziare la sanità a ristoro della ferita ancora aperta è evaporato per motivi di contesa politica assolutamente ingiustificata e intollerabile.

l'Italicum ha determinato un grande pasticcio. Noi abbiamo la necessità di non fare un salto indietro nel passato, a un sistema proporzionale che farebbe prevalere gli inciuci di palazzo rispetto alla volontà del voto e degli elettori. Su queste basi e con queste considerazioni, presidente Gentiloni Silveri, il Gruppo Conservatori e Riformisti non può accordare la fiducia al suo Governo. Ma noi le garantiamo rispetto, lealtà, coerenza e propositività. La nostra sarà una posizione rigorosa ma costruttiva, rispettosa del Paese ma anche del coraggio da lei dimostrato. Signor Presidente, l'auspicio è che il suo Governo voglia tornare a occuparsi dei problemi e delle emergenze del Paese e del popolo italiano dopo l'ebbrezza della insostenibile leggerezza della propaganda pseudoriformista. Grazie, e buon lavoro.

apprezziamo le sue parole, volte a richiamare al senso di responsabilità tutte le forze politiche, anche di opposizione, e non solo le forze di maggioranza che sostengono il suo Governo. Preliminarmente, esprimiamo la stima per la coerenza del suo predecessore che, pur avendo chiari numeri per continuare a governare, con un gesto eticamente nobile, raro nella politica dilagante dell'insulto e del tanto peggio tanto meglio, ha dato lezione di rispetto per le istituzioni, etica politica alla quale noi vogliamo continuare a credere e ispirarci. L'impegno, in questa fase delicata, deve essere quello di condurre i cittadini quanto prima al voto, attraverso un percorso condiviso e largo di scrittura delle nuove leggi elettorali. tale percorso venga rivolto anche alle forze politiche di opposizione. Noi, che non facciamo parte della maggioranza, ma siamo e restiamo forza di opposizione, coerentemente ai nostri principi liberali e riformisti di area di centrodestra, riteniamo doveroso collaborare alla scrittura e all'approvazione della riforma elettorale, così come, per gli stessi motivi, abbiamo sostenuto la riforma costituzionale. Solo scrivendo insieme le regole del gioco si può raggiungere la necessaria stabilità nel Paese ed assicurare con le prossime elezioni la piena governabilità. Quanti, dai banchi dell'opposizione, ora affermano di voler votare subito dimostrano di non avere davvero a cuore l'interesse dei cittadini, perché con il sistema attuale non vincerebbe nessuno e sarebbe necessario l'ennesimo inciucio per formare il futuro Governo. Forse è quello che vogliono, ma hanno anche la sfacciataggine di accusarla di essere un altro *Premier* non votato dal popolo, quando sono loro che, bocciando la riforma costituzionale, hanno impedito che il futuro Presidente lo sia. Contribuire a scrivere un nuovo sistema elettorale che garantisca un vincitore certo alle prossime elezioni, e quindi la governabilità, è un dovere di tutte le forze politiche, e del centrodestra *in primis*. E noi cercheremo di dare il nostro contributo in tal senso. Non voteremo contro la fiducia al suo Governo, che nasce con lo scopo fondamentale di affrontare la riforma elettorale. Non faremo opposizione acritica, ma con spirito propositivo e collaborativo siamo pronti ad assumere l'impegno di contribuire a svelenire il clima di ostilità e a dare il nostro apporto ai provvedimenti che saranno utili nell'interesse del Paese.

tra quelli che il suo predecessore, in più di un'occasione, chiamava i capponi, quelli che avrebbero fatto la brutta fine prima di Natale, quelli che stavano qua seduti in Aula

Ha ragione, Presidente, e hanno ragione anche gli osservatori parlamentari quando dicono che la nostra è una democrazia parlamentare e, di conseguenza, un Governo sta in carica se ha la fiducia di entrambe le Camere. È vero, ma è altrettanto vero che, visto che non siamo degli automi, un Governo deve capire quando è il momento di farsi da parte.

peste e corna dell'attuale Costituzione. E oggi voi giurate sulla Costituzione. Abbiamo ascoltato, Presidente, il suo intervento e la prima domanda che ci poniamo è questo non doveva essere un Governo per fare la riforma elettorale e poi andare al voto? Il suo programma di Governo mi sembra più quello che noi temevamo e quello che i cittadini temevano: un Governo a medio-lungo termine; un Governo che, se può, dura fino alla fine della legislatura. D'altronde, ad ascoltare gli elogi che sono arrivati da alcuni colleghi che hanno parlato prima di me - se dovessero andare a casa, ahimè,

scorso a dire «Io non penso alla poltrona» fu l'attuale ministro Fedeli, bravissima e stimatissima collega senatrice. Nell'enfasi e nella voglia di andare dietro ai deliri dell'ex Presidente del Consiglio, disse la stessa cosa, che bisognava andare a casa se avesse vinto il no. È stata premiata per la sua coerenza da senatrice e Vice Presidente del Senato a Ministro. Bella roba! Questo Governo è composto anche da chi penso all'attuale Ministro dell'interno - il 16 ottobre diceva a Reggio Calabria che l'immigrazione accelera lo sviluppo. Pensi lei agli italiani che in questo momento sono alla canna del gas, a quei milioni di italiani che non arrivano a fine mese e si sentono dire dall'attuale Ministro dell'interno che l'immigrazione accelererà lo sviluppo.

siete la continuità; voi continuate il vostro operato, quello che avete fatto fino ad ora; quello che avete fatto nei mille giorni in cui eravate a fianco dell'ex presidente Renzi. Mille giorni di disastri. E nell'enfasi in cui i colleghi si sono persino alzati in piedi dopo il suo intervento, ricordo zero influenza in politica estera. In politica estera non abbiamo contato niente - ahimè, Presidente - e forse è per questo che l'hanno messa lì: almeno non ha fatto danni. Dopo 148 voti a favore e zero contrari nelle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, spero che almeno lei possa fare quello che Renzi non ha fatto e che prometteva agli italiani di fare: un po' di dignità a livello europeo. 500.000 nuovi immigrati in mille giorni, come abbiamo detto prima, grazie al *tour operator* «Alfano&Co»; ce li hanno portati e - ahimè - ne porteranno ancora. Sono 208.000 gli italiani emigrati grazie alle vostre politiche economiche.

106 miliardi di nuovo debito pubblico: sono soldi degli italiani, sono i debiti che i nostri figli pagheranno perché voi avete fatto i fenomeni per 1.000 giorni. 130.000 risparmiatori sono stati truffati dalle banche degli amici, dei parenti, dei papà e di chissà chi, e che andrete avanti a tutelare; senza contare il 28 per cento degli italiani a rischio povertà e il fatto che l'anno scorso hanno chiuso 19.000 esercizi commerciali: 19.000 famiglie ridotte sul lastrico. Ma voi vedete la luce, Presidente. Voi vedete la luce. Una riforma al mese aveva promesso il suo predecessore. Spero che lei abbia almeno la decenza di non venirci a fare promesse da pulcinella come sono state fatte negli anni scorsi. Le ricordo la buona scuola:

Penso all'umiliazione delle Forze dell'ordine e del Corpo forestale dello Stato. Penso ai Vigili del fuoco precari. Tutti li chiamate eroi ma, quando i Vigili del fuoco precari hanno chiesto aiuto al vostro Governo, vi siete girati dall'altra parte. Voi siete tutto questo e siete anche tante di quelle cose che per motivi di tempo non sono riuscito a dire. Qualcuno dice che questo Governo serve - come ho detto prima - per fare la legge elettorale e andare al voto. La legge elettorale la fa il Parlamento, non il Governo. Non serviva questo Governo per fare la legge elettorale. Serve la volontà parlamentare per fare la legge elettorale il più velocemente possibile e per andare al voto ancora più velocemente. Quindi, vi sfidiamo: sfidiamo il partito della *cadrega*; sfidiamo tutti coloro che dicono di andare al voto, ma poi sono attaccati a quella che ognuno di noi ha dietro. Andiamo al voto il più velocemente possibile e confrontiamoci con gli elettori. Noi vogliamo votare, signor Presidente. Non vogliamo un altro Presidente del Consiglio che faccia il Renzi-*bis*.

proprio perché siete quello che eravate prima e non è cambiato niente e proprio perché - ahimè - farete quello che avete fatto prima, non meritate il nostro voto,

tra poco la fiducia e il mandato pieno. Le auguro un bel giorno. A noi senatori non c'è bisogno di fare l'augurio, perché il bel giorno non è un evento a venire, ma è la realtà dei fatti,

precedente Presidente del Consiglio che, da fenomeno qual era, era un po' un'eccezione, tutto era diventato eccezionale.

- in questo caso da parte del popolo italiano, che è il divieto a partecipare non alle manifestazioni sportive, ma alle sedute parlamentari - visto che, finalmente, non lo abbiamo né qui, né nell'altro ramo del Parlamento. ha chiesto come fece Renzi, promettendoci e quasi minacciandoci che quella sarebbe stata l'ultima volta, con un'esaltazione di sicumera che si avvitava - glielo dissi allora e lo ripeto adesso - con una certa particolare presuntuosa ambizione.

abbiamo avuto un Governo di piccoli accordi e la conseguenza è stata dividere oltremodo il Paese, di alimentare - l'ha detto lei - un'*excalation* verbale che ci ha dilaniato. La conseguenza è stata bloccare i processi decisionali, non fare riforme o farle così male da essere subito ampiamente bocciate dal pubblico e dalla critica: una legge sugli appalti illeggibile, quelle sulla pubblica amministrazione e sulle banche caducate dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato. E si trattava - diceva il Presidente del Consiglio di allora - della burocrazia, dei parrucconi, dei gufi, o sarebbe meglio parlare di un *ex* Presidente che era un giusto *mix* tra un apprendista stregone e un dilettante allo sbaraglio. la fiducia io, perché non condivido le sue idee su Stato e mercato, sulla perimetrazione dei diritti civili, sulla linea di equilibrio tra potere politico e organismo giudiziario. Ma condivido le sue idee su come il Governo debba incidere sulle riforme costituzionali e sulla legge elettorale. La legge elettorale è la legge - lo abbiamo detto in quest'Assemblea dalla nostra parte, quando non la votammo con quella fiducia

un Governo che brandiva lo scioglimento delle Camere per indurre il Parlamento alla morte lenta anziché al suicidio immediato. È stata fatta una legge elettorale con il voto di fiducia: orrore e ancora orrore. Abbiamo piegato, o meglio alla volontà del Governo. La legge che doveva attuare la Costituzione è stata votata a scatola chiusa solo perché il Governo la voleva; questo significa dare la fiducia sulle leggi. Non solo, la legge elettorale è stata fatta prima che vi fosse la nuova Costituzione, talché ora, senza quella nuova Costituzione, bocciata e strabocciata dal corpo elettorale, siamo senza legge elettorale. Lo avevamo detto, lo avevamo gridato in quest'Aula, ma abbiamo subìto la migliore delle prove di arroganza e presunzione. E quella legge, che avevamo detto essere incostituzionale, come ora dicono tutti, quella legge che Renzi diceva essere la più bella del mondo, che tutti ci avrebbero copiato, oggi è *tamquam non esset*. E come non ricordare una legge di bilancio piegata oltremodo alle occorrenze elettoralistiche, una legge già bocciata in Europa, della cui pesante eredità Ho già detto di forma e sostanza. Aggiungo che tra forma e sostanza c'è di mezzo la responsabilità, che è uno dei principi fondanti delle migliori democrazie. La responsabilità, soprattutto quando guidi il Governo e la macchina amministrativa, sta tra la forma che hai in mente di te stesso e la sostanza dell'azione del Presidente del Consiglio. L'ex Presidente del Consiglio è stato irresponsabile nel trascinare e piegare il bene degli italiani alla sua partita politica. Spero - e in parte sono convinto - che ella, signor presidente Gentiloni Silveri, non lo farà. Concludo, Presidente del Senato. Dicono i conservatori britannici, osservando la sequenza storica dei loro Governi e la loro durata, paragonandola a quella dei Governi laburisti, che è logico che vi sia stato nella storia britannica il doppio di Governi conservatori rispetto a quelli laburisti, perché ci vuole tempo per rimediare agli errori dei governi laburisti. Così chiedo a me stesso: quanto tempo ci vorrà per rimediare agli errori del Governo precedente? Certamente più tempo di quanto la residua durata della legislatura consenta a lei, presidente Gentiloni Silveri. Arriverà, quindi, a noi questa eredità, che sarà dura da ricevere. Purtroppo ci toccherà, ma ce ne assumeremo l'onere per il bene del Paese, pensando che di Governi come quello precedente l'Italia non ne debba subire per molto tempo. Presidente, signor Presidente del Consiglio, prima di tutto buon lavoro per il gravoso compito che l'attende. Credo che, nell'affrontare questo dibattito sulla fiducia al nuovo Governo, non si possa che partire da una constatazione: in dieci anni, per due volte consecutive, il popolo italiano ha bocciato le riforme costituzionali che abolivano il bicameralismo paritario e portavano a una semplificazione dell'*iter* legislativo, mettendoci al passo con le altre grandi democrazie. Il 4 dicembre scorso il *referendum* si è trasformato in uno *tsunami* che ha travolto il precedente Governo, perché il divario tra no e sì è stato vistoso e perché l'altissima partecipazione al voto ha conferito alla consultazione una formidabile valenza politica. Le conseguenze sono state inevitabili e il presidente Renzi ne ha preso correttamente atto, con un discorso da *leader* che sa assumersi le responsabilità. È proprio il concetto di *leadership* che va approfondito: Renzi, con la sua provvisoria uscita di scena, ha chiuso una lunga stagione politica imperniata proprio sulla preminenza dei *leader* nei confronti dei partiti e su partiti forgiati a immagine e somiglianza dei *leader*. Ora tutto cambia, e non gattopardescamente perché nulla cambi, ma perché lo ha voluto il popolo sovrano, che per paradosso, proprio nel momento in cui prevalgono l'antipolitica e le pulsioni antisistema, ha scelto di spingere il corso delle cose verso la restaurazione della vecchia politica. E dunque gli anni in cui si votava per i partiti o per le coalizioni - ma in realtà la sera delle elezioni si conosceva già chi sarebbe stato il capo del Governo - verranno soppiantati dal ritorno pieno, nella sostanza oltre che nella forma, ai riti della democrazia parlamentare. La modernità della politica richiede altro, ma oggi di fatto il Presidente del Consiglio non è più il *leader* assoluto del Governo, ma solo il *primus inter pares* nel Consiglio dei Ministri, ed è quello il luogo deputato a determinare in modo più collegiale di prima le decisioni politiche. Per questa ragione avevamo chiesto di sedervi. Questo Parlamento, nato senza maggioranza, si era dato una funzione costituente e ha fallito, perché la riforma costituzionale è stata respinta dal popolo e perché anche la legge elettorale maggioritaria, l'Italicum, il cui combinato disposto avrebbe garantito la governabilità ed è invece stato liquidato come una deriva autoritaria, è finita nel cestino. Il nostro Gruppo ha sostenuto con coerenza tutto il percorso riformatore, si è impegnato nel Paese, durante la lunghissima campagna referendaria, per sostenere le ragioni del sì è dunque stato compartecipe di una sconfitta. Del resto, anche il Governo a sua guida, signor Presidente, è in questo senso un Governo di sconfitti, partorito da una sconfitta. Ma non possiamo né vogliamo rinnegare il nostro contributo parlamentare a una grande scommessa sul futuro del Paese, che purtroppo si è rivelata perdente, anche perché, grazie ai nostri voti, negli anni scorsi sono state approvate in quest'Aula riforme importanti. Cito solo la più significativa, ossia la legge sulle unioni civili, che senza di noi non sarebbe mai passata. Lo abbiamo fatto per convinzione politica, stando fuori dal Governo Renzi, in diciassette lunghi mesi, mettendolo al riparo dalle insidiose divisioni nella maggioranza e garantendo non solo l'approvazione di decine di provvedimenti, ma la stessa funzionalità del Senato, con la tenuta del numero legale in Aula e nelle Commissioni. Questo senza mai nulla chiedere. Ma, nonostante tutto, la nostra generosità è stata direttamente proporzionale agli insulti che abbiamo ricevuto. Signor Presidente del Consiglio, mi scuso se ho fatto il riassunto delle puntate precedenti, ma davanti a lei, che ha definito il suo Governo come quello della responsabilità, ho il dovere di ricordare, per non fare torto alla verità, che i primi responsabili di questa legislatura siamo stati noi e che, quando si è aperta la crisi, abbiamo offerto la disponibilità a partecipare a pieno titolo all'azione di Governo. Sarebbe stato il coronamento di un percorso duro, tormentato e difficile, ma anche il raggiungimento di quella piena legittimazione politica di chi ha contribuito alla governabilità del Paese, in un momento storico in cui l'avanzata populista determinata dalla crisi economica richiede risposte forti e una migliore qualità della politica. Preoccupazioni più volte espresse dal presidente Mattarella, che ringraziamo per l'impeccabile ruolo di arbitro imparziale che ha svolto anche in questa circostanza. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*. Preoccupazioni che lei credo non abbia saputo cogliere appieno. Ma a lei, presidente Gentiloni Silveri, va ugualmente il nostro rispetto come Capo del Governo della Repubblica, anche se ci ha cortesemente chiuso la porta in faccia per ragioni presumo interne agli equilibri della sua maggioranza, col retropensiero di farci entrare magari in un momento successivo da qualche porta secondaria. Ma vede, questo è un Governo che avrebbe dovuto segnare una discontinuità rispetto al precedente, proprio per le circostanze in cui è nato; invece è la fotocopia quasi esatta del Governo Renzi senza Renzi. Questo è un Governo che avrebbe dovuto allargare la sua base parlamentare e ridurre le poltrone. Lei invece ha fatto il contrario, aumentando il numero dei Ministri. Ma siamo adulti e vaccinati e non inclini al risentimento e, dunque, non ci aggregheremo al coro degli urlatori da stadio, né ai fautori del «tanto peggio, tanto meglio», purtroppo oggi padroni della vastissima e insidiosa piazza del *web*, dove veicolano quotidianamente il loro odio, forti di un consenso popolare senza precedenti. Non è nel nostro DNA e non lo sarà mai. Semplicemente faremo opposizione al suo Governo, un'opposizione seria, rigorosa e mai sopra le righe, senza però alcuna indulgenza, sia che si tratti di provvedimenti che non ci convincono, sia che si tratti di quotidiane procedure parlamentari. «È la politica», diceva don Camillo, e lei la politica la conosce bene. In fisica, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Nella nostra visione politica questo automatismo non esiste. Esiste invece un principio molto più grande della fisica, che è quello della dignità politica, quella che lei, Presidente, non ci ha voluto riconoscere, sulla base di una *conventio ad excludendum* che ci consenta di non comprendere. La aspettiamo dunque al varco, presidente Gentiloni Silveri. Siamo convinti che la nascita del nuovo Governo sia necessaria, perché andare a votare a febbraio con due leggi elettorali diverse per Camera e Senato sarebbe stato irresponsabile e perché le emergenze del Paese vanno affrontate da un Esecutivo nella pienezza dei suoi poteri. C'è il dopo-terremoto; ci sono i conti correnti bancari dei risparmiatori da mettere in sicurezza; c'è l'emergenza immigrazione da governare, e spero che finalmente l'Italia riesca a far sentire la sua voce in Europa per modificare quel Regolamento di Dublino che ci costringe ad affrontare da soli le ondate migratorie come Paese di primo approdo. C'è la secolare questione del Sud, cui sono state fatte promesse mai mantenute. C'è, infine, l'esigenza di cui dovranno farsi carico Parlamento e Governo di varare leggi elettorali armoniche per Camera e Senato, perché è tornata la Prima Repubblica, ma non possiamo più permetterci la palude dei Governi instabili. Tutto spinge verso un ritorno al proporzionale, ma la nuova legge andrà ponderata con attenzione, dunque senza *Blitz* e senza fughe in avanti da parte di nessuno. Lei, Presidente, ha detto che il suo Governo durerà finché avrà la fiducia del Parlamento: frase lapalissiana, ma densa di significati politici per un Governo che sarebbe dovuto nascere solo per fare la legge elettorale. Tuttavia, gli impegni gravosi che la attendono avrebbero richiesto - questo parere - soprattutto qui al Senato, numeri certi per non correre il rischio di una navigazione da Governo balneare. Non sarà così, visto che noi la fiducia non possiamo dargliela e non gliela daremo per decisione convinta e autonoma del Gruppo: per intenderci,

strada. Concludo, Presidente, dicendo che questo è un Governo non all'altezza delle sfide che ha di fronte il Paese, perché ha una base politica e parlamentare troppo debole e precaria. Per questo annuncio che il nostro Gruppo non parteciperà al voto di fiducia. *(Applausi Signor Presidente, i senatori del Gruppo Per le Autonomie hanno condiviso e sostenuto la formazione del Governo Gentiloni Silveri, un Governo con pieni poteri,

e porti all'adozione di quei provvedimenti di riforma - dal processo penale alla legge sulla concorrenza - il cui *iter* è già stato avviato e che da tempo sono all'esame delle Camere. In ordine all'iniziativa del Governo, è evidente che il suo Esecutivo, signor Presidente del Consiglio, abbia priorità programmatiche che richiamano in primo luogo il ruolo dell'Italia in Europa, dalla legge di bilancio al sistema bancario, ma anche al terremoto e che giustamente ella ha definito con un riferimento esplicito alle emergenze sociali ed economiche del Paese; priorità che non sono soltanto in continuità

ha adoperato parole di grande equilibrio anche in merito alla questione della legge elettorale, in particolare quando ha affermato che occorre discontinuità nel dibattito pubblico. Ai Gruppi parlamentari,

ad assumere l'iniziativa sulla legge elettorale, perché è una nostra prerogativa alla quale non possiamo e non dobbiamo abdicare. Demandare la soluzione della questione della legge elettorale alla Consulta sarebbe devastante per l'immagine del Parlamento, perché sarebbe la conferma dell'incapacità della politica di decidere. È impensabile andare al voto con due leggi elettorali stravolte dalla Corte, con un Porcellum e un Italicum trasformati in Consultellum, ambedue di difficile attuazione per mancanza dell'intervento attuativo del legislatore. Tutti noi sappiamo che la sentenza della Corte, anche qualora cancellasse il ballottaggio e il premio di maggioranza, potrebbe essere non sufficiente per andare al voto con regole certe. Così come neppure il cosiddetto Consultellum è di per sé applicabile, perché restano aperti punti essenziali a iniziare dalla scelta del Parlamento sul sistema delle preferenze. Proprio coloro che invocano oggi, come anche in passato, le elezioni subito sarebbero i primi a incolpare questa maggioranza di aver causato un pasticcio Non è dunque, a nostro giudizio, credibile, né auspicabile, né sostenibile ipotizzare un Parlamento che si defili in attesa della sentenza della Corte costituzionale, dimostrando di non avere la volontà o la capacità di individuare un sistema elettorale condiviso. Il Gruppo delle Autonomie speciali, per quel che riguarda le leggi elettorali, ha indicato a lei, signor Presidente del Consiglio, l'esigenza fondamentale della conferma della riforma elettorale dei collegi

di passaggio della riforma, sia in caso contrario. In questo senso, siamo a posto. Siamo certi che il suo Governo garantirà anche una continuità dell'azione del precedente Governo Renzi con il quale abbiamo lavorato e collaborato molto bene anche nei rapporti con le autonomie; azione azione che ha portato a risultati estremamente positivi riducendo notevolmente il contenzioso davanti alla Corte costituzionale, esploso invece durante il Governo Monti. Siamo fiduciosi di poter portare a termine, con questo Governo, anche il lavoro già avviato negli ultimi anni, in particolare con il varo della norma di attuazione sull'amministrazione della giustizia per la Regione Trentino-Alto Adige ma anche per la Valle D'Aosta. Dovrà essere normata, finalmente, la cessazione degli accantonamenti illegittimamente disposti nel 2012, anche per tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. Noi, signor Presidente del Consiglio, siamo fiduciosi e certi di poter collaborare con lei in modo molto positivo e, per queste ragioni, il Gruppo per le Autonomie voterà la fiducia al suo Governo.

Sinistra Italiana non voterà la fiducia al suo Governo. Dopo il risultato referendario avevamo chiesto discontinuità, in modo chiaro e inequivocabile. Registriamo certamente un cambiamento dei toni che lei, Presidente, ha usato anche poco fa in quest'Aula, e un garbo istituzionale di cui non dubitavamo, conoscendola, e a cui eravamo disabituati dopo tre anni di vero e proprio bullismo esercitato dal suo predecessore nei confronti del Parlamento. Non possiamo che apprezzarlo, ma ciò non può bastare a noi e soprattutto ai quasi 20 milioni di italiani che il 4 dicembre hanno bocciato senza appello la vostra riforma costituzionale. Si è infatti risposto con una sorta di di Governo clone del Governo precedente e con la rivendicazione di tutto l'operato del Governo Renzi che, del resto, è lo stesso che chiede oggi la fiducia. Ma voi tutti sapete perfettamente che il no al *referendum* era in larghissima parte un no alle vostre politiche economiche, sociali e ambientali, era il rifiuto di tutte le riforme con cui il Governo Renzi, in tre anni, ha accresciuto le diseguaglianze sociali e ha falcidiato i diritti dei lavoratori e dei cittadini. È questa continuità che non possiamo in alcun modo accettare Presidente del Consiglio, anche nelle repliche, ha caparbiamente rivendicato, con il solito *mantra* dell'innovazione. Certo, è cambiato il Presidente del Consiglio. Matteo Renzi ha presentato dimissioni che erano in realtà un atto dovuto, se la dignità in politica ha ancora un senso, ma ha fatto capire a tutti, anche oltrepassando il confine della cortesia istituzionale, che a comandare e a decidere vuol essere sempre lui, tant'è vero che ha voluto mettere i suoi pretoriani a guardia del nuovo Esecutivo. La Ministra che aveva dato il suo nome alla riforma, dopo aver assicurato che se la riforma fosse stata bocciata avrebbe lasciato la politica, occupa in questo Governo una postazione molto importante e, oserei dire, strategica. Dopo annunci demagogici, non ha avuto la decenza politica di fare un passo indietro. L'ex sottosegretario Lotti, braccio destro del *Premier* uscente, viene promosso a ministro e mantiene, proprio con la Boschi, il potere di decidere nei prossimi mesi una quantità di nomine importantissime. Andarsene per finta e scrivere letterine su Facebook è facile, ma a rinunciare al potere reale Matteo Renzi, evidentemente, non ci pensa proprio. La stragrande maggioranza dei giovani ha votato no, non solo perché ha riscoperto fino in fondo il grande valore e l'orgoglio della nostra Costituzione, ma anche per bocciare il *jobs act*, che li condanna a una vita di precariato e di lavoro sottopagato e all'umiliazione dei *voucher*. Eppure, oggi oggi siamo chiamati a ridare la fiducia allo stesso Ministro del lavoro - sì, il Ministro dei *voucher* - come torna a chiedere la fiducia la stessa Ministra della pubblica amministrazione, che ha affrontato una riforma tra le più complesse, con l'intento solo di privatizzare i servizi pubblici locali, rovesciando la decisione presa dagli elettori con il *referendum* sull'acqua e sovvertendo il dettato costituzionale dell'imparzialità della pubblica amministrazione, tanto da arrivare a una clamorosa bocciatura da parte della Corte costituzionale. È cambiato solo il Ministro della pubblica istruzione: ci auguriamo che possa invertire la rotta disastrosa imboccata con la riforma chiamata, con sinistra ironia, buona scuola, ma ci speriamo poco. La verità è che in quei milioni di no al *referendum* c'è un grido di profonda sofferenza sociale, resa più estrema dalle riforme sbagliate del Governo Renzi. È una sofferenza dovuta all'assenza di lavoro, all'umiliazione del lavoro e dei lavoratori, all'insufficienza della sanità pubblica, che ogni anno ci regala milioni di persone che rinunciano a curarsi, alla povertà crescente, ma né il Governo né la maggioranza del PD, che di questo Governo è stato l'artefice, intendono ascoltare quel grido. Del Paese reale non avete capito niente. Per tre anni siete stati ubriacati dalla vostra stessa narrazione e ancora adesso, nonostante le pesanti smentite della realtà, continuate a non voler vedere e a non voler capire. Si chiede anche di concedere la fiducia a un Ministro di segnalarla. È una scelta incomprensibile e io direi irresponsabile, tanto più a fronte degli impegni internazionali di grande rilevanza che ci aspettano, la Presidenza di turno del G7 e il confronto nell'Unione europea su temi urgenti come l'immigrazione. Infine, ricordo la questione della legge elettorale. Speriamo sia definitivamente tramontata l'illusione di poter scrivere le regole del gioco a proprio uso e consumo. Serve una legge elettorale il più possibile condivisa, in linea con la Costituzione e che restituisca agli elettori il diritto di scegliere i propri rappresentanti e senza la distorsione della rappresentanza politica attraverso i premi truffa. Dopodiché, bisognerà andare immediatamente alle elezioni. Ci auguriamo con tutto il cuore che lei, Presidente del Consiglio, faccia davvero quel che ha promesso nel suo discorso e lasci al Parlamento tutta la libertà e l'agio necessari per mettere a punto una legge elettorale il più possibile condivisa, senza le incredibili forzature con cui fu imposto a colpi di voti di fiducia l'Italicum. Almeno questo segnale di discontinuità, Presidente, ce lo aspettiamo. Per il resto, però, questo Governo è un'offesa per gli elettori che il 4 dicembre hanno fatto sentire forte e chiara la propria voce. Il suo segno è dato dall'arroganza con cui un gruppo di potere decide di ignorare la volontà popolare. Può sembrare a voi una prova di forza. Invece è una prova di debolezza: questo Governo è un fortino assediato che prova disperatamente a blindarsi nella speranza di resistere e di passare la nottata. In questo disperato tentativo date ancora una volta prova della vostra totale irresponsabilità. Prima avete spaccato il Paese, cercando di imporre lo stravolgimento della Costituzione. Ora, dopo che il popolo italiano con il *referendum* ha dimostrato di avere ancora fiducia nella democrazia e speranza nella politica, sapete dare solo la risposta più brutale e sprezzante. A quei milioni di elettori state dicendo: «Tanto voi non contate niente». In omaggio all'ambizione smodata e alla sete di potere di un un piccolo gruppo di politici ambiziosi, rischiate così di distruggere la residua fiducia dei cittadini nella possibilità di cambiare le cose con il voto. Seminate distacco e rabbia. Quello che definite populismo è frutto della vostra irresponsabilità. Voglio solo ricordarvi che appena due giorni fa avete giurato solennemente di servire gli interessi del popolo italiano, non quelli di un gruppo di potere o di un segretario di partito. Lei, presidente Gentiloni Silveri, ha richiamato al rispetto delle istituzioni, ma, purtroppo, siete voi che ancora una volta dimostrate di non avere questo rispetto, innanzi tutto nei confronti della volontà del popolo sovrano. Per quanto riguarda noi di Sinistra Italiana, la valanga di no che ha difeso la Costituzione e sconfitto voi, che volevate stravolgerla, ci impegna oggi a dire no al suo Governo e a proseguire nella battaglia per cancellare le riforme che Renzi ha inflitto agli italiani, a partire dal *referendum* che toglierà di mezzo, a furor di popolo, il vergognoso *jobs act*, per costruire insieme ai tanti cittadini che hanno animato la battaglia per difendere la nostra Costituzione quel cambiamento vero che l'Italia si aspetta e in cui spera.

la presenza in quest'Aula di questo Governo è la risposta più eloquente ai tifosi del «tanto peggio tanto meglio», che nel nostro Paese sono sempre tanti, a quei profeti della sventura che, guidati da miopia politica, avrebbero voluto spingere l'Italia e gli italiani nel baratro di elezioni anticipate, dove dove l'assenza di una legge elettorale omogenea per Camera e Senato avrebbe consegnato il Paese all'ingovernabilità, mentre ci sono tantissime famiglie colpite dalla devastante sciagura del terremoto che attendono un impegno da parte di questo Parlamento e ci sono migliaia di famiglie che vedono i loro risparmi in bilico. Fortunatamente, oggi possiamo dire a tutte queste famiglie che un Governo politico, forte e saldo, ci sarà. Per questo risultato ringrazio per primo il presidente della Repubblica Mattarella, che con saggezza ha saputo guidare il Paese in questo difficile passaggio, richiamando tutti all'impegno di lavorare affinché il affinché il clima politico possa articolarsi e svolgersi con un rapporto dialettico, come è necessario per la nostra democrazia, ma sereno e costruttivo. Sbaglia chi pensa che questo Governo sia semplicemente un modo per evitare le urne o che sia la sala d'attesa per le elezioni. Chi oggi esprimerà il proprio voto di fiducia ha ben compreso il messaggio giunto dagli italiani il 4 dicembre. Le dimissioni del presidente Renzi rappresentano plasticamente la presa d'atto: un gesto coraggioso e coerente con quanto aveva dichiarato durante la campagna elettorale e che gli va riconosciuto con rispetto. Ma, all'indomani di un voto che ha diviso e lacerato profondamente il tessuto sociale e politico del nostro Paese, rifugiarsi nella corsa al voto sarebbe stato per questa classe politica, per questo Parlamento un pessimo segnale, quasi un'ammissione di incapacità, una resa. Vorrei ricordare a noi tutti che il secondo comma del primo articolo della nostra Costituzione recita che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti indicati dalla Costituzione. Ebbene, quelle forme e quei limiti siamo noi, tutti noi parlamentari a cui spetta il compito di garantire la governabilità. Gli italiani e tutti noi torneremo a votare, ma in uno scenario nel quale i fili del nostro tessuto sociale saranno finalmente riannodati, ritrovando quella necessaria serenità dopo una campagna referendaria divisiva e lacerante. Non dobbiamo dimenticare che c'è l'esigenza di armonizzare le due leggi elettorali della Camera e del Senato e che questo passaggio è indispensabile per andare a votare. In questo contesto, andare subito al voto avrebbe rischiato di lasciare il Paese in balia della confusione e con una sola certezza: l'assenza di un quadro politico, uscito dalle urne, chiaro, chiaro, che potesse rappresentare una seria e credibile proposta di Governo. Dinanzi a tutto ciò abbiamo ritenuto che fosse nostro compito assumere il peso di questa responsabilità, con convinzione, con impegno e soprattutto con speranza;

sanità pronta a governare l'innovazione, la valorizzazione della ricerca italiana, una grande attenzione alla fragilità del nostro territorio e importanti risultati nel campo della difesa. Vi è la speranza, è la speranza, signor Presidente, che alla fine potremo consegnare agli italiani un sistema Paese più capace di rispondere alla domanda di innovazione, di inclusione sociale e di governabilità.

non partecipiamo soltanto nella logica della responsabilità nazionale, ma in una visione di prospettiva politica. Si tratta per noi di un passaggio importante e nodale, non casuale, perché nuovamente a sostenere il peso di questo momento è la maggioranza che finora ha assicurato, responsabilmente, la governabilità di questo questo Paese. Spiace che l'appello che abbiamo rivolto ai partiti per un Governo di responsabilità nazionale sia stato seppellito dagli interessi particolari, a conferma che è sempre più diffusa tra le forze politiche e parlamentari la ricerca del consenso attraverso il populismo. Il voto di fiducia di oggi fa ulteriore chiarezza e disegna una maggioranza, un polo positivo che lavora per un'Italia migliore e che vuole guardare con fiducia al futuro, ma affrontando con serietà le emergenze presenti nel nostro Paese. A sua volta non riteniamo questo un Governo a termine o addirittura nato morto, come qualcuno si è affrettato a dichiarare. Non siamo nell'imminenza di elezioni; siamo piuttosto nell'imminenza della nascita di un Governo nel quale crediamo e sul quale puntiamo per continuare il buon lavoro finora portato avanti. Oggi Oggi nasce il governo Gentiloni Silveri e basta, e voglio dirlo chiaramente, signor Presidente, perché nessuno pensi che esista una spina da poter staccare quando si vuole, o di avere la *golden share* sulla vita dell'Esecutivo. Date di scadenza non ce ne sono: questo Governo andrà avanti fino a quando avrà i voti in Parlamento e quando avrà affrontato quelli che il presidente Mattarella ha indicato come adempimenti, impegni e scadenze, sia interne, sia europee sia internazionali. Questa è la rotta che dovremo seguire e sarà in Parlamento e non altrove che si deciderà il percorso di questo Esecutivo. Ricordo a tutti, infatti, che la nostra è una Repubblica parlamentare e non plebiscitaria e sono lieta che nel suo intervento, presidente Gentiloni Silveri, abbia voluto confermare la centralità del Parlamento la crisi di Governo non ha consentito di affrontare in quell'occasione. A tal proposito, infatti, sollecito l'Esecutivo ad intervenire rapidamente, così come celermente dovremo portare sostegno ai nostri concittadini colpiti dal terremoto, avviando la ricostruzione e continuando la lunga strada tracciata con il piano Casa Italia. Spetterà sempre a questo Governo prendere coscienza e parlare a quel 60 per cento che ha votato no e che ha espresso un disagio, al Sud, a quel ceto medio che più di tutti ha subìto il peso della crisi e dell'ondata della migrazione. Saluto con piacere la scelta del presidente Gentiloni Silveri di aver previsto un Ministro che si occuperà delle politiche del Mezzogiorno nella persona del professor De Vincenti.

il percorso di riforma della legge elettorale. È importante che la nuova legge nasca dal confronto tra le forze parlamentari, libere di individuare il sistema che meglio si adatti alla stagione che stiamo vivendo. Per questo ritengo che il percorso di revisione possa iniziare immediatamente, senza attendere la sentenza della Consulta, nella consapevolezza che con il voto del 4 dicembre si è conclusa la stagione maggioritaria del nostro Paese. È sempre più chiaro che il bipolarismo, che ha caratterizzato gli ultimi venti anni della nostra storia, ha lasciato il passo a un tripolarismo e di questo la nuova legge elettorale non potrà non prendere atto. di una legge «contro» qualcuno o qualcosa, ma di una legge «per»: per governare, per dare stabilità al Paese, per garantire agli italiani piena rappresentanza nelle Aule parlamentari. L'esperienza del recente passato guidi la nostra azione. Per questo rivolgo un appello a chi oggi darà il suo voto a questo Governo e a chi non lo darà, affinché si lavori insieme per dare nel più breve tempo possibile agli italiani una buona legge elettorale.

dovremo resistere alle sirene del populismo e di chi farà di tutto per portare la rotta del Governo sugli scogli. Ma siatene certi, in questa maggioranza, nei volti e negli occhi di ogni singolo senatore, senatore, troverete quel sostegno e, soprattutto, quelle motivazioni per andare avanti, quelle che oggi sono alla base del nostro convinto voto di fiducia. *(Applausi

oggi stiamo vivendo un momento drammatico nella vita del nostro Paese e onestamente in quest'Assemblea sto avendo un'allucinazione, perché davanti a me vedo le solite facce. Sono poche, perché sono già spariti tutti, neanche il tempo di ascoltare le dichiarazioni di voto: questo è il rispetto che hanno per il Parlamento.

a quel Governo e quella maggioranza, che l'hanno portata avanti paralizzando il Parlamento per due anni e lasciando sui banchi del Governo tutte le emergenze di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non lo abbiamo detto il nostro ex *Premier* che da quella riforma sarebbero dipese le sorti politiche del Governo! Ma oggi ritroviamo qui la maggior parte degli stessi Ministri. E non venite a dirci che Renzi se n'è andato, perché Renzi non

Luca Lotti, al quale vengono date le deleghe per lo sport e che mantiene la delega all'editoria. Editoria e informazione, cittadini!

in una fase iniziale a suon di continue forzature e ricatti è stato il suo secondo, grande e grave errore. Strappare al centrodestra pezzetti e pezzettini, immaginando che fossero politicamente rappresentativi, mentre il baricentro rimaneva saldamente ancorato alla figura di Silvio Berlusconi, è stato un ulteriore azzardo pagato molto caro.

a tutto questo non sono convinto sia una risposta sufficiente dare il titolo a un nuovo Ministero. Questo è il giudizio che ricaviamo dal voto al *referendum* del 4 dicembre, e credo che non possa che essere condiviso dalle tante persone perbene ed intellettualmente

dei rappresentanti nelle istituzioni, prendendo ad esempio l'esperienza francese dei repubblicani di Fillon, Juppé e Sarkozy di pochi giorni fa. Occorrono regole certe e riconosciute da tutti i contendenti, con il supporto dell'apparato statale e un risultato accettato senza esitazioni da tutte le parti in gioco. Leggi vanno a completamento della regola democratica per eccellenza che siamo chiamati a scrivere, rappresentata ovviamente dalla legge elettorale. Se è vero, come credo, che la prossima legislatura dovrà essere costituente, questo ci obbliga a elaborare una nuova legge elettorale che sia in grado di interpretare in maniera più fedele possibile la volontà dell'elettorato, pur garantendo la governabilità. Solo così, con una rappresentanza pienamente legittima, dovuta a una forte base proporzionale della legge elettorale, il prossimo Parlamento sarà legittimato a modificare la nostra Costituzione nel nome del popolo italiano.

Mi auguro che il nostro Primo ministro abbia un approccio differente rispetto a quello avuto negli ultimi tre anni da Matteo Renzi: meno provocazioni estemporanee e più preparazione, meno politica muscolare e più continuità e vigore nella difesa del ruolo e delle esigenze nazionali. Solo così, in Europa, si può arrivare a risultati concreti. Gli argomenti del prossimo Consiglio europeo mi sembrano molto importanti e strategici per il nostro Paese: immigrazione, sicurezza, economia, giovani (compreso il tema del contrasto alla disoccupazione giovanile) e relazioni internazionali. Su questi argomenti ci aspettiamo un'azione efficace che il precedente Governo non è stato in grado di svolgere: una stringente lotta contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo per interrompere quella che è ormai rimasta l'unica e più pericolosa grande rotta migratoria; una vera difesa dei confini europei; una politica economica che segni finalmente la discontinuità, abbandonando l'austerità in favore di un nuovo modello di sviluppo; un piano europeo per facilitare l'accesso al lavoro giovanile, la definizione di una politica di difesa comune comune e, infine, di una politica europea unitaria che affronti *in primis* la questione turca, la crisi ucraina e il tema delle sanzioni alla Russia, ma che soprattutto ridoni al vecchio Continente il rilievo e il ruolo che gli competono. Ho apprezzato il riferimento fatto da lei, Presidente, nei sui interventi di ieri alla Camera e di oggi al Senato al quadro di relazioni tra le grandi potenze (Stati Uniti, Russia, Europa) che si sta definendo intorno alla crisi siriana. È proprio in riferimento a scenari come questo, mutevoli e in divenire, che l'Europa e l'Italia hanno il dovere di tornare tra gli attori principali, in uno scacchiere internazionale sempre più caratterizzato dalla tensione tra Stati Uniti e Russia e dalla frammentazione in più fronti del conflitto interno al mondo islamico tra sunniti e sciiti, dalla Siria all'Iraq (ha dimenticato lo Yemen), fino al tema curdo, il più grande popolo senza uno Stato. Due notizie hanno contrassegnato queste ultime ore: la liberazione di Aleppo e la rioccupazione di Palmira da parte del Daesh. Palmira, come sapete, è l'esempio di città romana meglio conservata al mondo e mi auguro che tra qualche ora non dovremo dire «era». Aleppo è una delle città più antiche della storia, rappresenta un grande esempio di convivenza tra popoli (arabi, armeni, curdi, circassi, turchi) e religioni, con una delle maggiori comunità cristiane del mondo arabo (circa 300.000 di diverse confessioni religiose), che ne hanno fatto una capitale culturale ed economica, riferimento dell'intera area, con una storia ininterrotta di cinquemila anni, messa in pericolo da gruppi armati di miliziani jihadisti ai quali la comunità internazionale ha voluto dare lo *status* di ribelli. È la nostra storia, la nostra cultura e l'Europa non può continuare a starsene ai margini. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Forza Italia non può dare fiducia al quarto Governo non eletto dal popolo italiano, ma ci auguriamo che in Parlamento, in questa Assemblea, si approvino velocemente regole certe, in grado di assicurare che la volontà popolare sia di nuovo rispettata. Signor Presidente, le senatrici e i senatori del Partito Democratico voteranno la fiducia al Governo dell'onorevole Gentiloni non soltanto per la stima e la considerazione che nutrono nei suoi confronti, ma anche per precise e decisive ragioni politiche. Tutti i senatori sanno che il Governo Renzi, poche ore prima delle dimissioni, proprio in quest'Aula, aveva ricevuto un ampio voto di fiducia, che avrebbe dovuto essere interpretato come fattore di continuità fino al completamento della legislatura. Viceversa, come aveva annunciato con un bel discorso dopo l'esito del *referendum* e proprio in ragione di quel risultato, il presidente Renzi ha rassegnato le dimissioni: una decisione impeccabile, a mio avviso, per il rispetto dovuto a un risultato che ha visto bocciare dal popolo il provvedimento cardine della legislatura. Ho letto le dimissioni di Matteo Renzi come un'assunzione di sua personale responsabilità

sarà necessario fare, anche per rispondere a tanta smemoratezza che sta segnando il dibattito politico e che è emersa sgradevolmente anche oggi in quest'Aula. Consentitemi solo di formulare a Matteo Renzi i miei più sinceri auguri per il suo futuro personale e politico in una nuova stagione di riforme utili all'Italia. Osservo che senza le sue politiche e le innumerevoli misure sull'economia, il lavoro, la scuola, la giustizia e la cultura non avremmo i tanti dati che testimoniano in modo inequivoco una stabile inversione di tendenza, l'uscita dalla recessione e la ripresa dell'occupazione. Venivamo da una situazione molto negativa e i risultati sono ancora insufficienti, ma oggi, senza quelle misure, saremmo a commentare dati molto diversi, se non opposti. Come sappiamo, abbiamo solo iniziato il processo di uscita da una crisi insieme economica e politica, sociale e istituzionale, che sarà ancora lunga e che non riguarda solo l'Italia, ma l'intera Europa, dalla Francia alla Gran Bretagna, dalla Spagna alla Grecia, che investe sia il Nord che il Sud, sia l'Est che l'Ovest del nostro Continente. Il lavoro di risanamento del nostro Paese deve, quindi, continuare le basi ci sono. Il presidente Gentiloni Silveri ha tutto l'equilibrio e l'esperienza necessari per guidare il Governo fino all'appuntamento delle elezioni che il Parlamento e le forze politiche chiedono vengano celebrate in tempi brevi, con una legge elettorale omogenea

Onorevole Gentiloni, lei presiede un Governo che è stato definito in vari modi; per le condizioni in cui il Governo nasce, preferisco anch'io chiamarlo Governo di responsabilità nazionale. L'orizzonte limitato e la prossima scadenza elettorale accrescono e rendono più impegnative le sue responsabilità. Nei suoi interventi, ieri alla Camera e oggi qui in Senato, c'è un punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea: mi riferisco al suo annuncio dell'impegno del Governo in materia sociale e sul terreno dei diritti. C'è oggi in Europa, e purtroppo anche in Italia, una seria e grave questione sociale che pesa sui giovani, sulle persone più anziane, sul Mezzogiorno, sulle periferie urbane, sui cittadini più in difficoltà, su una povertà sempre più ampia. Poco fa ne ha parlato con grande efficacia il senatore Tronti. Non è nelle possibilità di un Governo cui è dato un tempo definito risolvere questioni di dimensioni gigantesche, che hanno avuto origine molti decenni fa e che sono andate seriamente aggravandosi, non solo per un contesto sempre più difficile, ma anche per nostre incapacità. Il Governo Gentiloni Silveri può però avviare le soluzioni, metterle a fuoco, sollecitare le iniziative, può mostrare con la sua politica che il Paese è sensibile verso realtà in crisi che meritano dal Parlamento e dal Governo un'attenzione speciale e misure all'altezza dei bisogni. Presidente Gentiloni Silveri, molto presto lei rappresenterà l'Italia in importanti appuntamenti internazionali, dovrà provvedere alle urgenze del dopo terremoto e far fronte all'emergenza della crisi bancaria. In questi impegni e in molti altri, lei sarà sostenuto dalla maggioranza che è emersa anche in questo dibattito e della quale i senatori del Partito Democratico sono e saranno parte convinta e determinante. Vengo quindi a qualche considerazione più politica sulla difficile fase nella quale il Governo inizia il suo cammino. Il contesto politico nel quale oggi ci troviamo presenta una profonda e vistosa crisi della democrazia in gran parte delle Nazioni dell'Occidente. Facciamo attenzione a non sottovalutare questo delicatissimo aspetto della nostra convivenza: la democrazia è la cifra principale della nostra civiltà, la radice delle nostre libertà. Ovunque, anche in Italia, la democrazia è stata conquistata con fatica, con il lavoro ed anche con il sangue; evitiamo di difenderla soltanto con le parole. Perdere la democrazia o anche soltanto indebolirla indebolirla per gli egoismi, per la frantumazione degli interessi e per una cecità che ci fa ignorare il contesto mondiale in cui ci muoviamo sarebbe un delitto imperdonabile. All'interno di questo quadro generale, vanno valutati gli interessi e le prospettive dell'Italia. Il risultato chiaro ed esplicito di un *referendum*, che tutti debbono accettare con lealtà (a partire da chi in Parlamento ha votato a favore della riforma), ha lasciato insoluto il grande problema dell'adeguamento del nostro sistema istituzionale alle esigenze dei cambiamenti radicali del nostro tempo e alla necessità di mettere il nostro Paese in grado di reggere la dura competizione internazionale con la quale quotidianamente dobbiamo fare i conti. Il tutto in coincidenza con la gravissima crisi istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea che, andando nella direzione opposta a quella federale indicata da Altiero Spinelli, oggi rischia la disgregazione. Sono queste condizioni complessive e la consapevolezza dello stato generale dei problemi ad aver spinto il Partito Democratico a sollecitare la formazione di un Governo sostenuto dalla più larga parte delle forze politiche presenti in Parlamento, un Governo che accompagnasse il lavoro di armonizzazione delle leggi elettorali di Camera e Senato e portasse, subito dopo, il Paese al voto. a larga base parlamentare nasceva dalla convinzione che, pur nelle diversità, anche profonde, che segnano le forze politiche di maggioranza e di opposizione, le condizioni dell'Italia e la limitata durata del Governo rendessero molto utile una sia pur breve forma istituzionale di coesione nazionale. Purtroppo una campagna elettorale che in più occasioni ha largamente oltrepassato i limiti di un ordinato confronto ha deteriorato i rapporti politici e ha impedito che quella iniziativa venisse intesa nel suo corretto significato e avesse un seguito positivo. Resta immutata - e dobbiamo farcene tutti carico - la necessità di abbassare i toni del dibattito politico e mostrare agli italiani un Parlamento meno rissoso e meno strumentalmente diviso. C'è troppa volgarità in giro, travestita da una certa politica, travestita da un certo giornalismo, travestita da una certa satira. È nostro dovere mostrare al Paese un Parlamento dove la lotta politica sappia riconoscere i confini del confronto civile. Lo dico con molta cortesia, prima di tutto a lei, senatrice Montevecchi, che oggi con le sue parole smodate e in molti punti infondate, con i suoi cartelli non ha certo dato un bello spettacolo di serietà politica. *(Applausi Sono queste le precondizioni che hanno portato all'indicazione dell'onorevole Gentiloni Silveri da parte del Capo dello Stato e alla successiva formazione del suo Governo. Una scelta saggia, quella del nostro Presidente, che garantisce la continuità di una politica estera, che è fattore decisivo per la stabilità del Paese, e assicura una presenza leale nei confronti dell'Unione europea, ma che, nel solco del Governo Renzi, è anche molto esigente in materia di politiche di sviluppo e di occupazione, di gestione delle migrazioni, di una sempre più vigorosa maturazione del processo di integrazione politica dell'Europa. All'onorevole Gentiloni Silveri, che ringraziamo per il servizio che si appresta a svolgere per il nostro Paese, vogliamo fare i nostri migliori auguri di buon lavoro, ben sapendo che il successo del suo Governo serve all'Italia e non alla maggioranza che lo sostiene, ma anche che le sue difficoltà sarebbero di ben poca utilità all'opposizione e farebbero molto male all'Italia.

Signor Presidente del Consiglio, riconosco come il suo sia un Governo necessario. Le forze politiche hanno infatti il dovere di corrispondere, già in questa legislatura, alle ragioni di un voto referendario così indicativo della volontà della Nazione, cercando con buona volontà un comune denominatore sulle regole e i criteri della rappresentanza in una democrazia che dobbiamo volere più inclusiva. Le società comprensibilmente non vogliono essere governate da minoranze organizzate. La stessa stabilità che queste possono garantire sulla base di premi elettorali smodati viene poi messa in discussione direttamente dal popolo. Al contempo, tuttavia, lei si pone in continuità con la precedente esperienza di Governo tra diversi, la quale da tempo ha esaurito le ragioni emergenziali su cui era opportunamente nata e che, per quanto mi riguarda, non può avere prospettiva alcuna. Penso che, alla base di ogni azione pubblica, vadano riproposti quei principi della tradizione nazionale che la sinistra vecchia come quella nuova mettono quotidianamente in discussione: la vita, la famiglia naturale, la libertà educativa. Tanto esprimerò un giudizio sui singoli provvedimenti libero e responsabile, quanto parteciperò alla ricostruzione di una cultura e di un'offerta politica conservatrice, liberale e popolare, come tale rigorosamente alternativa alla sinistra. Per queste ragioni non parteciperò all'espressione del voto di fiducia. Signor Presidente, ho vissuto un sogno: quello di contribuire a poter cambiare il nostro Paese, come fu nel 2006. Il popolo ha deciso e noi dobbiamo prenderne atto. Ormai ogni ipotesi di riforma è archiviata nell'agenda politica. Si volevano meno parlamentari e oggi abbiamo più Ministri. Questo Governo nasce su basi che non posso e non voglio condividere: un assestamento degli equilibri interni al partito di maggioranza in un'ottica congressuale e una conservazione di poltrone utile a gestire un potere autoreferenziale. Il risultato sarà che i cittadini si rivolgeranno sempre di più verso una deriva populista e velleitaria. Mi dispiace, presidente Gentiloni, perché ho per lei un grande rispetto e ho avuto modo di apprezzarla come ottimo Ministro degli affari A titolo personale annuncio quindi il mio voto di sfiducia a questo Governo, un voto che per tanti non ha alcuna importanza ma che per la mia coscienza di uomo libero ne ha tantissima.

votazione nominale con appello sulla mozione di fiducia n. 703, presentata dai senatori Zanda, Bianconi e Zeller:

Grazie,

e non vengono risparmiati i bambini. *(Brusio).* Vi chiedo un po' di attenzione perché è una strage che si sta compiendo da molti mesi. Negli ultimi due giorni, però, vi è stata una recrudescenza e le organizzazioni umanitarie hanno registrato un aumento dei bombardamenti. Si vedono immagini strazianti che fanno capire che possono essere state usate armi chimiche, vietatissime, come il fosforo bianco e il cloro. Abbiamo notizie di circa un centinaio di bambini, assediati in un edificio nella parte est della città, nella quale sono in atto scontri pesantissimi. Sono fonti verificate, non stiamo parlando di ipotesi: ci sono - ripeto - molte fonti verificate e non è possibile equivocare. È una situazione drammatica in cui i civili, i bambini, sanno che la prossima bomba o il prossimo proiettile alla testa potrebbe essere per loro; stanno molto peggio dei topi in gabbia, stanno attendendo una fine atroce e non si sta facendo quanto si dovrebbe per fermare questo massacro. Qui i diritti umani vengono calpestati e cancellati in nome di ragioni militari e politiche che, sappiamo, sono paraventi perché dietro, come sempre, ci sono le ragioni economiche di uno scacchiere geopolitico internazionale in cui c'è bisogno di gas, di petrolio, di materie prime. Sulla base di questo continuano i massacri. Si parla già di 300.000 vite umane: una media città. 300.000 vite umane già scomparse, un esodo di milioni di persone.

Ecco, Aleppo è la punta dell'*iceberg* di centinaia di situazioni di stragi e di illegalità profondissima. Il mio vuol essere un appello a tutte